con l'emendamento 5.103 si interviene

nel 2006 e nel 2009 con l'estensione dei casi di arresto obbligatorio in flagranza:

ossia gli atti sessuali con minorenni. Su questo tema c'è stata anche, nei mesi scorsi, forte polemica.

la violenza si ritiene presunta. Ovviamente ci sono dei casi di minore gravità, sia negli atti di violenza sessuale,

bene.

possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. Noi riteniamo che per i soggetti condannati per questo tipo

«la partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 4,

è prevista dall'ordinamento penitenziario esclusivamente per i reati di sequestro di persona. mentre, sotto il profilo della gravità del reato, è prevista la possibilità di non avere, se non dopo quel determinato numero di anni, l'ammissione ai benefici, trattamenti psicologici, rieducazione, eccetera, è giusto prevedere anche un divieto di concessione dei benefici, se non dopo gli anni previsti (i due terzi della pena)

Signora Presidente, gli argomenti che ha svolto il sottosegretario Caliendo mi portano ad un dubbio. Quindi, prima di commettere - o indurre l'Assemblea a commettere - un errore, preferisco in questo momento ritirare l'emendamento. Ci sarà un'altra

parere favorevole

proprio per nascondersi rispetto a questi atti di violenza nei confronti dei minori. È passato il principio per cui nell'ambito familiare sarà punita qualsiasi violenza contro i più deboli; non solo, è passato anche il principio per cui chi ha dei minori a carico per l'esercizio di una professione o di un'arte sarà punito se il minore diventerà merce ed oggetto di violenza. Con questo articolo abbiamo introdotto nuove modifiche al codice penale che riconoscono nuovi reati e inaspriscono ulteriormente le pene per chi li commette.

vorrei fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia, con qualche considerazione su questa Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, che è il primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i bambini diventano reati. reati. Oltre ai reati più comunemente diffusi in questo campo la Convenzione disciplina anche i casi di adescamento attraverso Internet e di turismo sessuale. La Convenzione - questa è la particolarità - delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre correre e di insegnare loro a proteggersi; stabilisce programmi di supporto per le vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono e via Internet. Certo è che con la diffusione e lo sviluppo di Internet si è assistito alla presenza di una nuova dimensione organizzata della pedofilia, che è in fase di incremento quantitativo. Se il *web* abbia poi effettivamente aumentato il numero dei pedofili «attivi» è difficile da dimostrare. Quello che è certo è che, di fatto, la Rete ha reso maggiormente fruibile la pedopornografia e ha consentito ai pedofili di aggregarsi in comunità, il che di per sé già già rappresenta un fattore di rischio in più. Sulla Rete si può trovare una serie di siti pedofili che non contengono materiale pedopornografico, ma che compiono una vera e propria apologia e sostituiscono precedenti forme di espressione sottoculturale, reperibili con grande difficoltà prima dell'avvento di Internet. L'attività investigativa nel corso del periodo 1998-2005 ha registrato un costante e significativo aumento. I dati disponibili mostrano abbastanza chiaramente il crescente impegno degli investigatori nel contrasto al fenomeno. Un ruolo altrettanto importante è stato svolto dagli esperti della polizia postale e delle comunicazioni, i quali rilevano come le violenze avvengano soprattutto tra le tra le mura domestiche e non riguardano solo le famiglie degradate, ma tutte le classi sociali e tutte le categorie di professionisti e che gli abusanti si avvicinano ai bambini gradualmente e in modo subdolo. Evidentemente, le caratteristiche che emergono dall'analisi dei dati riferiti alle segnalazioni all'autorità giudiziaria, non possono essere rappresentative dell'intero universo. Le informazioni a nostra disposizione fino ad ora rispondono alle specifiche finalità istituzionali delle amministrazioni che le raccolgono. In realtà, lo studio del fenomeno dello sfruttamento ed abuso sessuale dei minori nella sua dimensione quantitativa non è facile. Il fenomeno stesso, infatti, presenta contorni non perfettamente definiti: gran parte di episodi di abuso sui minori non viene infatti denunciata per molteplici ragioni e per ciò sfugge a qualsiasi rilevazione statistica. L'obiettivo dell'organismo costituito presso la

nella maggior parte dei casi, a siti pedopornografici. Il dato più significativo riguarda però le segnalazioni di *file sharing* che sono cresciute dell'85,4 per cento passando da 165 a 306.

I dati quindi invitano ad una riflessione attenta sull'evoluzione continua della pedofilia in Internet e sul ruolo che ciascun soggetto (legislatore, istituzioni, polizia, *provider*, associazioni specializzate) è chiamato a svolgere con responsabilità e particolare attenzione per evitare ritardi o indecisioni i cui costi per le bambini ed i bambini coinvolti sono ancora tanto alti da risultare realmente Si stima che un sito pedopornografico registri da un minimo di 7.000 ad un massimo di 20.000 contatti al giorno; l'aumento di questo tipo di siti tra il 1997 ed il 2005 è stato del 1.500 per per cento, mentre solo nell'ultimo anno è stato del 60 per cento. Anche i dati più aggiornati riferiti al 2009 continuano a mostrarci un fenomeno di proporzioni veramente allarmanti, soprattutto alla luce delle considerazioni precedenti circa il fatto che i reati scoperti ed inseriti nelle statistiche rappresentano solo la punta dell'*iceberg*. Sono 570 i siti dai contenuti illeciti finiti nella *black list* da quando è stata istituita tre anni fa. Una volta entrati nella *black list* i siti diventano inaccessibili dall'Italia e dagli altri Paesi che aderiscono al sistema di condivisione e scambio delle *black list*.

televisivi americani. La pedofilia è, dopo la droga, la principale preoccupazione dei genitori. È un timore

primo dei quali è non dare confidenza agli estranei e poi chiedere immediatamente aiuto e non rivelare informazioni private come *e-mail* o numero di telefono. Un genitore su tre dice di non sapere ancora come comportarsi e a chi rivolgersi nel caso i figli fossero vittime di abusi; inoltre, per circa il 60 per cento dei genitori i figli sono poco informati sui rischi della pedofilia. Ogni anno sono 41.000 i nuovi casi di violenza sui minori. Per questo dobbiamo impedire tali aberrazioni con ogni mezzo, perché la tutela dei bambini, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico e spirituale, deve costituire il nostro obiettivo primario, rispetto al quale non possiamo permetterci alcuna esitazione. Per il senso di responsabilità che tutti dobbiamo avere

per l'Italia su questo provvedimento, che rappresenta senza dubbio un passo importante nella lotta a quello che può essere considerato il reato più aberrante: la violenza sui minori.

Il mondo, evolvendosi nel corso di questa strada per migliorare le condizioni di vita, di esistenza, ha scoperto nuovi fronti criminali prima quasi inesistenti. Uno dei settori più aggredibili e più indifesi è proprio quello dei minori. Non è un bel progresso quello della nostra civiltà nel momento in cui

dobbiamo sempre aggiungere nuovi reati, perché la fantasia dell'uomo è fertile e genera sempre nuove condotte criminali. Non è un bel progresso, il nostro, però riusciamo ancora a difenderci, ad individuare, in un'analisi che abbiamo fatto nel corso dei lavori parlamentari, in uno scambio di opinioni e attraverso

come fosse necessario irrobustire le leggi, prevedendo sanzioni verso nuovi reati,

o l'adescamento dei minori via Internet: crimini dei tempi moderni. Noi diamo delle risposte non solo ratificando la Convenzione di Lanzarote, ma anche adeguando il nostro ordinamento interno. Penso si sia fatto un buon lavoro.

di un progresso che ci fa scoprire che la nostra società diventa sempre più vulnerabile e necessita sempre di più di risposte penalistiche.

che si possa dire ai criminali, ai pedofili, agli adescatori, a coloro

Le puntuali e tecniche modifiche del codice penale e di procedura penale a mio avviso possono essere riassunte e ricomprese in tre profili. primo attiene al fatto che si recepisce uno strumento internazionale, uno strumento che vuole sancire un livello comune di lotta ad un fenomeno così esecrabile e che oggi, nel villaggio globale, sottolinea che l'internazionalità è il modo con cui questo problema deve essere affrontato. Ne consegue un altro profilo, che deriva direttamente da questo: particolare attenzione nel provvedimento è messa sul profilo della Rete,

non rende più l'idea del qui e là. Là è tutto: accanto a noi c'è sempre un bambino che ha bisogno di un'attenzione,

in modo che i bambini possano continuare a sognare senza dover incontrare troppi uomini neri sulla rete, compia un'azione particolarmente buona. In un giorno in cui qualche dichiarazione, forse non del tutto felice, sulle attività dei senatori viene mandata alle stampe, io ritengo che oggi il Senato possa raccogliere per sé un motivo di fierezza.*(Applausi

parlando ai colleghi, io vorrei trasmettere uno scatto di orgoglio, proprio perché, in ambito di sfruttamento sessuale minorile, il nostro Paese, rispetto a tutti gli altri Paesi europei, è considerato fra i più avanzati, avendo già recepito nel proprio ordinamento nuove norme in ambito di nuove tipologie di reato proprio in materia di abusi sessuali. anche dire che l'Italia ha recepito per prima la Convenzione sulla protezione dei bambini dagli abusi sessuali, approvata dal Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 e che noi, lo stesso anno, il 7 novembre, abbiamo sottoscritto. La Convenzione di cui stiamo parlando adesso, la Convenzione di Lanzarote, è il primo strumento a livello internazionale che considera reati tutte le diverse forme di abuso sessuale in danno di bambini e di adolescenti.

le proposte che prevedono il nuovo reato di *grooming*, ossia di manipolazione psicologica dei minori; che hanno previsto la creazione di unità investigative specializzate, chiaramente sotto copertura, per indagare sulla pedopornografia; che hanno previsto il rafforzamento della cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di questi reati; la creazione di un fondo per le vittime degli abusi; l'introduzione del reato di corruzione di minore; l'allontanamento del reo dal nucleo familiare, qualora ne fosse un membro; l'identificazione dei minori ritratti su materiale pedopornografico; la creazione di osservatori nazionali; la previsione di altre misure a protezione del minore. Oggi, nel nostro ordinamento, con la legge di recepimento, introduciamo altri aspetti del diritto di carattere più procedurale e penale, come il raddoppio dei termini di prescrizione se l'interessato è un minore di età inferiore a 14 anni; l'inasprimento delle pene per l'associazione a delinquere finalizzata a reati sessuali,

Vorrei aggiungere che, come Lega Nord, ci siamo trovati quasi sempre in prima fila per combattere questo fenomeno. Vorrei ricordare che la settimana scorsa abbiamo depositato un'ulteriore proposta di legge sui reati efferati o, meglio, quelli realizzati con particolare crudeltà,

niente benefici e niente sconti di pena. Abbiamo introdotto nell'ordinamento penitenziario un articolo 41-*ter* che va a sommarsi al 41-*bis*, meglio conosciuto come carcere duro per i mafiosi ancora pericolosi. Ricordiamo anche l'azione di questo Governo: infiniti sono stati i decreti sicurezza del nostro ministro Maroni; inoltre, su questa materia è stato introdotto il reato di *stalking*, ossia per ogni tipo di molestia, come pure

In Commissione si è ritenuto collegialmente di dover inasprire le pene per tutti i reati a sfondo sessuale, e ci siamo trovati sostanzialmente tutti d'accordo: c'è stata molta unità su questo

soltanto per l'atto sessuale, in caso di lieve entità, mentre questo non è previsto per la violenza. Cosa stava a significare? Che se due minori, ad esempio un sedicenne e una tredicenne, venivano colti da un pubblico ufficiale

in procinto di essere arrestato, avesse dichiarato: no, sto violentando questa ragazza, il pubblico ufficiale non avrebbe potuto più fare nulla. Chiaramente era un un palese errore, una contraddizione, una disarmonia. Pensiamo di aggiustare il danno combinato, anche perché volevamo evitare che dei ragazzini finissero in carcere loro malgrado; ma ahimè, come capita spesso, la questione viene strumentalizzata e alcuni colleghi fanno addirittura girare su quelle catene comunicative simili a *blog* che i presentatori di questa sistemazione - se mi si passa il termine - ossia i senatori Bricolo, Divina, Mazzatorta e Gasparri che avevano firmato l'emendamento, messi così alla gogna - sarebbero stati i protettori dei pedofili. figuriamoci! Siamo qui per fare leggi - lo stiamo dimostrando - per perseguirli, per far sì che le pene siano certe, per condannarli; figuriamoci se siamo qui per difendere i pedofili.

Noi comunque siamo convinti che siano i fatti e le azioni a rendere poi giustizia. Proprio oggi, ahimè, non è stato accolto - noi pensiamo per disarmonia con il testo - un emendamento mio e del collega Mazzatorta che prevedeva addirittura l'introduzione di un reato definito turismo sessuale, proprio perché conosciamo i meccanismi che alimentano il fenomeno. Non è passato in questa occasione: ci sarà il contenitore più adatto per riarmonizzare il tutto.

che preventive che dovranno coinvolgere una pluralità di soggetti: pensiamo alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle famiglie, alla scuola

Questo ha comportato che un provvedimento licenziato dalla 2a e dalla 3a Commissione sia stato, peraltro non per nostra volontà, un po' abbandonato, anche se non del tutto, perché molti colleghi sono stati in Aula. signora Presidente e colleghi, vorrei sottolineare che oggi è un giorno molto importante, perché concludiamo in Senato l'*iter* di un provvedimento parlamentare che riguarda lo sfruttamento e l'abuso sessuale sui minori grazie ad interventi condivisi di opposizione e maggioranza, allarga lo sguardo anche ai maltrattamenti in ambito familiare e di convivenze equiparabili. Mi riferisco alla nuova formulazione della norma prevista dall'articolo 572 del codice penale, che si viene così ad aggiungere alla norma fortemente voluta dal Partito Democratico sullo *stalking* che è già stata approvata in questa legislatura. Ho già detto questa mattina quanto sia importante la nuova formulazione dell'articolo 572 del codice penale, ma intendo insistere su questo argomento, perché lo ritengo proprio un punto qualificante del percorso che è stato svolto in Senato e che ci consentirà di combattere più efficacemente le violenze in famiglia contro i minori e le donne. Detto questo, gli abusi contro i minori sono tra i fatti più riprovevoli e tra le forme di violenza peggiori. Privano infatti il minore della libertà e della dignità e ne pregiudicano, spesso irrimediabilmente, il percorso di vita e lo sviluppo della personalità. Un bambino molestato o abusato difficilmente avrà un'autostima; forse non sarà mai un cittadino con la stessa grinta di un altro, con la stessa voglia di conquistarsi un giusto ruolo nella società, con la capacità di vivere autonomamente un protagonismo sociale. Con il disegno di legge che ci accingiamo a varare, cercheremo - mi auguro - di arginare questo terribile fenomeno. Le molestie, le violenze e gli abusi sui minori sono fatti gravi, spesso di difficile emersione ed accertamento, soprattutto perché molte volte si realizzano in contesti familiari o di convivenze, in circuiti educativi o comunque in ambienti che dovrebbero, per definizione, ritenersi protetti. La Convenzione adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa a Lanzarote, sottoscritta il 7 novembre del 2007 dall'Italia, si inserisce nella serie di numerosi strumenti internazionali a tutela dei minori, primo tra tutti la Convenzione di New York del 1989. Agiamo nell'ambito della tutela dei diritti umani. La Convenzione di Lanzarote affronta in via sistematica le tematiche dello sfruttamento e dell'abuso sessuale con una serie di misure, come la protezione in via anticipata del minore, la costruzione di una barriera di prevenzione, l'istituzione di autorità specializzate, gli interventi per prevenire e reprimere tutte le forme di sfruttamento sessuale, per diffondere la percezione e la consapevolezza della problematica, soprattutto nei circuiti e tra le persone che hanno relazioni e contatti con i minori nel campo dell'educazione, della salute, della protezione sociale e degli organismi di polizia addetti alla prevenzione, alle investigazioni e alla repressione.

Il testo su cui preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, ha avuto uno sviluppo parlamentare complesso, perché trae origine da varie iniziative parlamentari, caratterizzate tutte da un comune denominatore: l'individuazione di misure effettive di tutela dei diritti fondamentali dei minori rivolte al contrasto dello sfruttamento sessuale e pedopornografico in qualsiasi forma realizzato. In Senato, dopo il grande impegno della Camera, si è pervenuti ad un testo unificato, ulteriormente discusso e perfezionato con il contributo delle opposizioni, grazie al lavoro eccellente svolto dalla relatrice, senatrice Allegrini. Difatti sono state aggiunte molte norme importanti di adeguamento dell'ordinamento interno. La linea ispiratrice di questo importante provvedimento legislativo, che per quanto riguarda l'Italia si inserisce in un contesto normativo già attento alla garanzia dell'integrità psicofisica dei minori, è quella di predisporre strumenti normativi adeguati per combattere le forme più subdole di violenza e abuso contro i minori. I dati dell'UNICEF ci sono noti: due milioni di bambini sono utilizzati ogni anno nell'industria del sesso; sulla rete Internet sono veicolate più di un milione di immagini di bambini abusati di questi solo 20.000 sono stati identificati, gli altri sono anonimi, probabilmente continueranno a subire abusi e forse non saranno mai identificati. A questa piaga sociale si tenta di dare una risposta con la nuova formulazione dei reati di adescamento di minori per scopi sessuali e di pedofilia e pedopornografia culturale, che ricomprendono condotte poste in essere anche con i mezzi di comunicazione tecnologicamente più avanzati. Si è data specifica attuazione così all'articolo 23 della Convenzione di Lanzarote, offrendo strumenti effettivi che consentono un intervento anticipato agli organi di polizia per impedire comportamenti propedeutici

e organizzazione a fini di profitto. Si è previsto un particolare rigore nell'applicazione delle pene accessorie derivanti dalle condanne e dal patteggiamento, così come alla confisca del profitto anche per equivalente derivante dalla riprovevole attività illecita di sfruttamento sessuale di minori. È giusto d'altra parte affermare che, se sono coinvolti minori, è necessario creare una rete adeguata di protezione e quindi sanzionare tutti i comportamenti di abuso sessuale che intervengono su persone fragili, immature, particolarmente suggestionabili e adescabili. Per questo si è reso necessario ed opportuno intervenire anche sul piano delle misure cautelari e, in particolare, con misure rimesse al giudice per vietare l'avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati da minori minori e nella materia della confisca penale obbligatoria, che costituisce un ulteriore elemento di prevenzione oltre che di repressione e di effettivo soddisfacimento dei danni. Ne è derivato complessivamente un confronto parlamentare, alla Camera e poi al Senato in Commissione giustizia e in Commissione affari esteri, che ha portato a norme ampiamente condivise. Ricordo che alla Camera si è intervenuti sul gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito delle persone offese minori vittime di violenza sessuale o di gruppo, di pedopornografia e di sfruttamento sessuale in genere e al Senato - come dicevo inizialmente - sono state introdotte tante nuove norme importanti e si è giunti finalmente a modificare il testo dell'articolo 572 del codice penale. L'impegno comune è stato quello di introdurre disposizioni più stringenti. Ovviamente non manca la consapevolezza che il provvedimento in discussione costituisce solo una parte importante di un percorso che deve essere arricchito da interventi che mirino ad isolare i fattori di disagio culturale e sociale. e sociale. Occorre, quindi, una politica che non tenda soltanto alla repressione penale e all'inasprimento sanzionatorio, ma che valorizzi come elemento di prevenzione fondamentale la formazione degli operatori della scuola, dei centri sportivi e culturali, delle forze dell'ordine e della magistratura e nel sostegno alle famiglie per dare finalmente attuazione al dettato dell'articolo 2 della Costituzione, perché quelle formazioni sociali

ed è soddisfatto del lavoro che trasversalmente si è riusciti a portare avanti in una materia così delicata.

sta portando ancora una volta alla ribalta l'orrendo fenomeno della violenza nei confronti dei bambini e degli adolescenti. Questi drammi, spesso confinati nelle mura domestiche, si tramutano altrettanto spesso in tragedia. Ci sono altri drammi che restano confinati nel silenzio e nella psiche delle piccole vittime che non riescono, che non possono reagire e che sono, a loro volta, tragedie infinite per chi le subisce. I bambini e i ragazzi sono ancora troppo spesso vittime indifese di azioni odiose, perpetrate da parte di adulti senza scrupoli, azioni che purtroppo, come più volte sottolineato anche in questa sede, condizionano per sempre il loro equilibrio psicofisico. Il riscatto di questi bambini e adolescenti violati è difficile perché l'umiliazione, l'introiezione del dolore e della propria dignità umiliata

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare, la ratifica della Convenzione di Lanzarote, rappresenta un fondamentale strumento internazionale - e questa è una cosa importantissima importantissima - per la tutela e la difesa dei minori contro le violenze e i soprusi commessi nei loro confronti in ogni situazione e ambito, anche in quello che dovrebbe essere per loro più sicuro, cioè la famiglia. L'obiettivo della Convenzione è costruire un percorso condiviso, di forte contrasto a ogni abuso nell'ambito, come si diceva, della tutela dei diritti umani, fermo restando che ogni Stato può continuare a predisporre ed emanare ulteriori misure, se vogliamo ancora più restrittive. È proprio questa la scelta fatta dal Parlamento italiano, impegnato in un'attenta azione assolutamente trasversale, Siamo orgogliosi del comportamento del nostro Paese che, come ben detto dalla collega Serafini e dal collega Divina, è all'avanguardia nell'azione di tutela verso i minori. Il nostro Paese non è mai stato a guardare - lo ricordo anche io perché già nel 1996 fu approvata la legge recante norme contro la violenza sessuale che ha inserito, per la prima volta, i crimini sessuali nell'ambito dei delitti contro la persona e non più contro la moralità pubblica e il buoncostume. Nel 1998 si fece un ulteriore passo avanti con la legge n. 269 recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che ha introdotto le nuove fattispecie di reato relative allo sfruttamento sessuale dei minori, con particolare attenzione alla prostituzione e alla pornografia minorile. Ricordo poi, colleghi, la recente legge del 2006 n. 38 recante questa disposizione in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, che ha operato sul piano dell'inasprimento delle pene detentive e sul contrasto dei reati di pedopornografia sulla rete Internet. In maniera, lo ribadisco, assolutamente trasversale il Parlamento ha deciso di attuare la Convenzione inserendo ulteriori adeguamenti, ovvero modificando il codice penale e il codice di procedura penale e inserendo norme diverse come, ad esempio, le misure di prevenzione e l'ordinamento penitenziario, con la finalità di garantire ai minori con ogni mezzo possibile il diritto a crescere senza abusi e senza violenze, trasformando i reati nei loro confronti finalmente in reati penali. La pedofilia, quindi, è una questione penale, un fenomeno criminale che indigna le coscienze e che deve essere contrastato attraverso l'efficace azione legislativa. Ancora prima, la pedofilia è una questione culturale, nel senso che per combatterla è necessario sensibilizzare la coscienza collettiva, la coscienza di tutta la società, perché si tratta di un crimine abominevole, inaccettabile, di fronte al quale nessuno può chiudere gli occhi e nessuno può far finta di niente. Se è necessaria la pena, tutti noi sappiamo che ancora più importante è un'efficace azione preventiva: se si arriva, infatti, ad applicare una pena vuol dire che un danno irreparabile è stato commesso e una o più vite sono state rovinate per sempre. Ecco perché, nonostante l'introduzione di norme di grande rilievo, finalizzate a garantire una tutela più pregnante alla dignità e alla stessa integrità psicofisica dei minori, sono emerse esigenze ulteriori di cui il Parlamento si è fatto carico proprio con il provvedimento che stiamo per votare. Oltre ai reati più comunemente diffusi in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), l'accordo disciplina anche, ad esempio, i casi di *grooming* (adescamento attraverso Internet) e trasforma in reato penale le pratiche inaccettabili di mutilazione degli organi genitali femminili, fino a prevedere la perdita della potestà del genitore. Finalmente! Data la natura sempre più transnazionale di tali reati e l'uso sempre maggiore delle nuove tecnologie, prima fra tutte Internet, le disposizioni dell'Accordo sono orientate a rafforzare la cooperazione fra i Paesi, soprattutto in termini investigativi. Non ci sono dubbi che la libertà di comunicazione sia sacrosanta, ma nasce la necessità per il legislatore di predisporre mezzi di controllo a tutela dei più piccoli, per prevenire ed evitare che le innovazioni tecnologiche possano diventare lo strumento per la diffusione e l'espansione di crimini odiosi come la pedofilia. In questo - e mi associo alle dichiarazioni della collega Serafini l'azione della polizia postale è determinante, anche per bloccare i reati di apologia della pedofilia commessi da coloro che usano la rete per disquisire tranquillamente di pedofilia. Il Senato ha apportato alcune sostanziali modifiche al testo approvato dalla Camera, che a nostro avviso rendono più incisive, se possibile, le finalità e l'obiettivo cardine di questo provvedimento. Mi riferisco, ad esempio, alla sostituzione del concetto di pedofilia culturale con quello di istigazione alla pedofilia, perché, come bene diceva la relatrice, senatrice Allegrini, nulla di culturale può essere associato al concetto di pedofilia. È stato poi introdotto il trattamento psicoterapeutico; è stato accolto l'emendamento del senatore Li Gotti e di altri senatori del Partito Democratico, che ha riscritto l'articolo 572 del codice penale sui maltrattamenti in famiglia, che riguardano finalmente anche le donne e i soggetti più deboli all'interno della famiglia,

è una bella pagina parlamentare, quella che stiamo scrivendo oggi. Con l'auspicio che, tornando alla Camera, questo provvedimento veda la conclusione del suo *iter* e possa entrare in vigore al più presto, instaurando così un patto sociale forte e coraggioso, perché la questione infanzia diventi un impegno e una sfida di tutti i Paesi, ringrazio innanzitutto per il sostegno e la collaborazione il Governo - nella persona del sottosegretario Caliendo

bene.

tenuto in 5a Commissione in relazione alla riforma della *governance* di politica economica che è in atto in Europa. È evidente a tutti che la la crisi economica che abbiamo subito nei mesi scorsi ha comportato una ovvia necessità di maggiore coordinamento e di modifiche delle procedure di *governance* a livello europeo. Parallelamente, ha fatto emergere le debolezze strutturali molto rilevanti nei meccanismi di sorveglianza esistenti; così come è emersa è emersa la necessità di integrare gli indicatori tipici di analisi della affidabilità delle finanze pubbliche con altri indicatori. Sulla base di queste considerazioni, bisogna anche tenere conto dell'approvazione del cosiddetto semestre europeo, quindi di un ciclo di procedure che impongono, da un lato, un insieme

insieme di meccanismi per migliorare la sorveglianza degli indicatori economici di bilancio dei singoli Stati. Prima di entrare nel dettaglio della riforma, bisogna tener conto

da un lato, da parte della Commissione europea, dall'altro - da parte dei Governi e, per la precisione, della cosiddetta *task force* che ha come rappresentante Van Rompuy - che hanno sugli argomenti che andiamo ad affrontare delle visioni spesso contrastanti. Per quello che riguarda il nostro modo di agire, è interessante capire verso quali posizioni si andrà a finire, in particolare su tre temi, che andiamo ad affrontare velocemente: la spesa pubblica, la spesa pubblica, il debito pubblico e le sanzioni. Sappiamo tutti che per governare queste due dimensioni, in particolare il debito e la spesa pubblica, si fa riferimento al Patto di stabilità e di crescita. Per quanto riguarda il Patto di stabilità e di crescita emerge la necessità a livello europeo di rivedere la *governance* generale, pervenendo ad un contenimento della spesa pubblica, da un lato, e alla riduzione del debito, dall'altro; quindi, intervenendo preventivamente sulla dinamica e l'evoluzione della spesa pubblica e, *a posteriori*, in azioni correttive di riduzione del debito pubblico. Emergono già le principali divergenze tra l'impostazione della Commissione e quella, invece, dei Governi, rappresentata dalla posizione della *task* *force* e di Van Rompuy. Per la spesa pubblica, per esempio, la Commissione prevede un tasso di crescita che dovrebbe essere inferiore al tasso di crescita del PIL a medio termine, definito come prudente, a meno che l'eccedenza non sia coperta da misure discrezionali sul lato delle entrate. Cerchiamo di tradurre questa definizione in qualcosa di più comprensibile

l'impatto che queste nuove norme che verranno decise possono avere sui margini di azione del nostro Governo e del nostro Parlamento. L'altro tema su cui vi è una certa divergenza riguarda il debito. Per il debito la Commissione prevede un meccanismo automatico e una riduzione definita quantitativamente in un ventesimo.

quantitativa precisa, ma in ogni caso anche la loro posizione va nel verso di una riduzione, da esplicitarsi poi in maniera corretta e chiara.

dibattito, sulla possibilità di fallimento del debito sovrano, ricordando la figura di Marco Minghetti, il Presidente del Consiglio di fine '800 sotto la cui Presidenza, per la prima e unica volta, il nostro Paese ha raggiunto il pareggio di bilancio. I dati che ci siamo detti impongono che, in futuro, noi dovremo necessariamente arrivare a questa condizione, cioè al pareggio di bilancio e al *surplus*. Ilterzo tema su cui vi è una divergenza interessante tra le posizioni della Commissione e quelle dei Governi riguarda le sanzioni, sanzioni, che sono molto onerose: si parla della costituzione di depositi fruttiferi in casodi sanzioni *ex ante* e non fruttiferi per le sanzioni*ex post*; in ogni caso si tratta di sanzioni molto onerose.

di sanzioni, ma con una procedura più graduale e con la possibilità da parte dei Governi stessi di intervenire in questa fase, evitando le sanzioni con una votazione qualificata. Passo ora ad un altro tema, che, però, è assolutamente rilevante per quanto ci concerne. Abbiamo appena riformato le procedure di bilancio con la legge

sarà necessario pervenire ad una modifica della legge di contabilità, non solo nella tempistica, ma anche nei contenuti dei documenti di programmazione economico-finanziaria, per renderli aderenti a questa nuova modalità di determinazione dei dei bilanci dei singoli Stati, però coordinati a livello europeo. Passando ad un altro tema, quello della cosiddetta sorveglianza macroeconomica, abbiamo fatto riferimento all'inizio della relazione al fatto che in futuro non si terrà conto unicamente di indicatori di bilancio tradizionali (ricordiamo il deficit e il debito pubblico al 60 per cento, giusto per rammentare gli indicatori tradizionali cui si fa riferimento), ma questi andranno integrati con altri indicatori di carattere macroeconomico che specificano meglio la situazione dei singoli Stati aderenti all'euro (fatto di assoluto interesse). Facciamo qualche esempio di nuovi indicatori che potranno diventare parte di questo *set* di indicatori dell'efficienza nella gestione dei singoli Stati. Per quanto riguarda gli indicatori di bilancio, ad esempio, si potrà considerare anche la quota del debito in scadenza nell'anno per valutare appunto la capacità di gestire l'indebitamento a breve; e ancora, sempre per quanto riguarda il rischio di bilancio, il *gap* dell'avanzo primario, tema essenziale per poter poi pervenire al pareggio di bilancio e quindi alla riduzione del debito. Per quello che riguarda il nostro Paese sono poi molto importanti gli indicatori di rischio macrofinanziario, che possono andare a integrare le valutazioni delle singole Nazioni. Si parla, per esempio, del saldo delle partite correnti (giustamente, visto che abbiamo un tasso di cambio fisso all'interno dell'euro; però, il saldo delle partite correnti, di fatto, approssima il tasso di cambio reale), del debito del settore privato (che è evidente indicatore della solvibilità a medio e lungo termine delle singole Nazioni: e fortunatamente, questo per noi è un fattore positivo, chiaramente sempre in relazione alle altre Nazioni europee), e ancora, della quota del settore immobiliare rispetto al PIL. per la Spagna avrebbe comportato valutazioni differenti. La Spagna, prima di entrare nella crisi attuale, aveva indicatori di bilancio pubblico assolutamente di livello, positivi, però chi avrebbe mai detto cinque, sei o dieci anni fa che la Spagna non era messa bene? E chi avrebbe dato peso ad un indicatore come quello della quota del settore immobiliare sul PIL? tutti sono concordi nel considerare questo un fatto rilevante ma, all'epoca, di sicuro nessuno lo avrebbe preso in considerazione (figuriamoci per comminare eventuali sanzioni). considerazioni solo per esemplificare il dibattito che si sta innescando su questi indicatori aggiuntivi e l'impatto che possono avere per le singole Nazioni.

addirittura, che Francia e Germania hanno messo nero su bianco nella loro intesa comune, che si possa pervenire ad opzioni concrete quali la sospensione del diritto di voto per le Nazioni ampiamente indipendenti rispetto ai *set* di parametri che verranno definiti. Ovvio che una modifica del genere è molto pesante e determina modifiche dei Trattati, cosa al di là da venire e non certo semplice, però la dice lunga sull'impatto di queste discussioni che vengono svolte a livello di *governance* europee sui margini di azione delle singole Nazioni. Insomma, la consapevolezza del processo in atto di devoluzione dei poteri di bilancio dalle singole Nazioni all'Unione europea dovrebbe diventare patrimonio comune di tutti i senatori. A mio modesto avviso, ciò faciliterebbe molto anche il dibattito, che spesso si in maniera molto settoriale, e anche un po' provinciale, sui singoli comparti dicendo che non si può ridurre questa spesa o quell'altra, mentre avremo di fronte la necessità di realizzare una riduzione della spesa molto, molto cospicua negli anni a venire, per non parlare della rivoluzione relativa alla riduzione del debito.

colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la crisi che ha investito l'Europa ed il resto del mondo ha gettato le basi per una *governance* economica europea ed ha ed ha attivato un percorso virtuoso di convergenza dei principi e delle regole per una migliore convivenza economica dei Paesi europei. Si tratta, a nostro avviso, di un percorso innanzitutto politico, politico, ma anche di procedure, che deve saper coniugare democrazia e responsabilità, che altro non sono che i pilastri della democrazia partecipata richiamata dal Trattato di Lisbona per un migliore funzionamento delle istituzioni europee e nazionali allo scopo di migliorarne incisività. Parliamo, quindi, di percorsi che, per raggiungere gli obiettivi, devono prevedere il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, a partire dal Parlamento. a partire dal Parlamento. Qui si apre la prima vera discrepanza tra la visione intergovernativa, che, pur avendo dato miseri frutti, risulta essere ancora la visione del Governo italiano, e la visione comunitaria che può garantire di più e meglio legittimità democratica, fiducia dei cittadini nelle istituzioni ed efficacia del risultato. Ad oggi, non risulta che il Governo abbia aperto un confronto su questo processo con il Parlamento e nemmeno assicurato il necessario e corretto flusso di informazione. ricordare, signora Presidente, che le carenze nell'organizzazione dei lavori del Senato ci ha portato oggi nella Commissione politiche dell'Unione europea a vivere una situazione di totale confusione generata dalla necessità di adempiere alle nuove procedure di partecipazione nel processo decisionale europeo, da una parte, in particolare per quanto riguarda i cinque provvedimenti già all'esame delle Commissioni di merito e della Commissione politiche dell'Unione europea per la valutazione di sussidiarietà e proporzionalità, e la necessità, tutta politica, di segnalare anche attraverso l'odierna risoluzione la particolare attenzione e preoccupazione del Parlamento rispetto alla riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani cui verranno assunte decisioni di rilevante importanza relativamente alla necessità di rafforzare il Patto di stabilità e crescita. A stigmatizzare questo contesto, bene si presta l'affermazione del presidente Van Rompuy nel suo intervento alla riunione della COSAC (Conferenza degli organi dei Parlamenti nazionali specializzati negli affari comunitari) in cui ha affermato che sempre di più c'è bisogno di pensare in modo globale ed europeo. Ora - purtroppo, sta diventando un'abitudine - l'Italia non si presenta nella migliore delle condizioni. In particolare, per quanto riguarda il debito pubblico e, in generale, per l'assenza di riforme che dovrebbero consentire al nostro Paese il superamento di una condizione di fragilità, come Come è già stato detto dal relatore, senatore Garavaglia, se l'obiettivo europeo è il coordinamento delle politiche fiscali e macroeconomiche, allora serve una conoscenza dettagliata delle misure di politica fiscale e di programmazione economica che gli Stati membri intendono attuare nel successivo esercizio finanziario. Ma il cosiddetto semestre europeo non corrisponde alla tempistica di programmazione prevista dalla legge italiana di contabilità e ciò potrebbe creare problemi di credibilità ed efficacia degli impegni assunti. Per garantire il maggior coordinamento delle politiche fiscali europee ed evitare le tensioni politiche e finanziarie degli scorsi mesi, il Consiglio propone una riforma della tempistica, con l'intenzione di esprimere una valutazione *ex ante* rispetto alle politiche fiscali nazionali. Se da un lato questa impostazione rappresenta un passo in avanti verso una trasparenza e un coordinamento maggiori a livello europeo delle politiche nazionali, dall'altro, almeno nel nostro Paese, pone problemi di compatibilità tra la tempistica dell'esame tecnico della Commissione europea e quella della programmazione economica interna. In altre parole, secondo quanto previsto dall'attuale legge di contabilità e quanto proposto dal Consiglio Ecofin, ad aprile il Governo italiano fornisce a Bruxelles indicazioni su misure di politica economica che verranno approvate dal Parlamento solo ad ottobre, dando luogo a quei problemi di credibilità ed efficacia degli impegni presi. La nuova versione delle linee guida introduce una sostanziale novità nella struttura dei patti di stabilità e crescita: il cosiddetto semestre europeo. le informazioni richieste dalle nuove linee guida non prevedono sostanziali novità rispetto al contenuto dei documenti esistenti. La Relazione unificata sull'economia e la finanzia il primo documento rilasciato dal Governo nel ciclo di bilancio previsto dalla legge n. 196 del 2009, riporta già alcune informazioni richieste dalle nuove linee guida. Oggi, però, la Relazione unificata sull'economia e la finanza viene semplicemente trasmessa al Parlamento a titolo informativo, aggiornamento sulla situazione delle finanze pubbliche. Va da sé che nel nuovo schema la Relazione dovrebbe cambiare il suo *status* ed assumere le caratteristiche dell'attuale Decisione di finanza pubblica; in questo modo il Programma di stabilità e convergenza presentato in sede europea conterrebbe conterrebbe gli obiettivi programmatici fissati dal Governo e discussi e approvati dal Parlamento, vincolando tanto l'organo legislativo quanto l'Esecutivo. A partire da ciò e mettendo in fila tempi e strumenti, diventa evidente allora come la disposizione europea sia in controtendenza rispetto all'orientamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica pubblica italiana: mentre la prima anticipa ad aprile alcuni degli elementi contenuti nella Decisione di finanza pubblica, la seconda opera nella direzione opposta, spostando la presentazione della Decisione di finanza pubblica da giugno a settembre. Se poi guardiamo al periodo di vigenza della legge n. 468 del 1978, che prevedeva il termine di presentazione della Relazione unificata sull'economia e la finanza per il 28 febbraio, troviamo una ulteriore conferma in tal senso: la presentazione effettiva del documento viene a cadere nella seconda metà del mese di marzo. Sarebbe così sufficiente anticipare il termine di presentazione indicato nella legge di contabilità e finanza pubblica. II maggior coinvolgimento del Parlamento nella identificazione delle intenzioni di politica fiscale rende necessaria una modifica allo schema previsto dalla legge n. Sarebbe quindi opportuno prevedere l'istituzione di una apposita sessione parlamentare dedicata proprio alla discussione ed alla definizione delle intenzioni di politica fiscale da sottoporre successivamente alla Commissione europea. Solo una maggiore armonizzazione tra l'impianto normativo nazionale e quello europeo potrà rendere la vigilanza fiscale prevista dal semestre europeo veramente efficace. al fine di intervenire efficacemente sugli Stati membri che violino le nuove regole, con la proposta di regolamento sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio si stabiliscono sanzioni finanziarie progressive. Per quanto riguarda la parte preventiva, deviazioni significative comporterebbero, a carico dello Stato membro interessato, l'obbligo di costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2 per per quanto riguarda la parte correttiva, il rispetto della normativa è garantito analogamente dall'apertura di un deposito infruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL al momento dell'apertura di una procedura di disavanzo eccessivo. Il deposito può essere convertito in ammenda in caso di non osservanza e la sanzione può essere ulteriormente inasprita in caso di persistente inosservanza, arrivando perfino, come propone la *task force* del Consiglio europeo, alla sospensione del diritto di voto in Consiglio. Sempre la *task force* suggerisce, come elemento essenziale per garantire un corretto funzionamento nella gestione delle finanze pubbliche, la creazione di organi indipendenti che forniscano l'analisi delle previsioni di bilancio nazionale predisposte dal Governo; in questo senso sarebbe auspicabile il ruolo autonomo del Parlamento, anche per assicurare controllo e trasparenza. Siamo allo stadio del *work in progress*, una fase decisiva per definire criteri e procedure atte a garantire la stabilità dell'eurozona, una fase che rischia di essere molto penalizzante per l'Italia che non riesce ad allineare le proprie procedure interne, neanche quelle minime di recepimento, rendendole compatibili con l'impianto europeo ed efficaci non solo per migliorare la credibilità del nostro Paese in Europa, ma anche per assicurare un ruolo decisivo, per dare un contributo alla *governance* economica europea e, allo stesso tempo, per rendere sostenibile per il Paese questa nuova ondata di rigore. Non è una problematica inerente solo ai trattati perché, come ha dimostrato Maastricht, in una situazione difficile, anche se non come quella attuale, decisivo è il ruolo ed il profilo che i Governi nazionali scelgono di assumere. Bisognerebbe piuttosto richiamare alla memoria e alla realtà, lo sforzo di coesione nazionale oltre che sociale ed economica, che l'Italia fu in grado di compiere in quella circostanza. Infatti, l'Italia si trova ad un bivio drammatico, tra necessità di contenimento del debito e necessità di sostenere la crescita. Politiche fiscali e contenimento del debito da soli non saranno in grado né di far uscire l'Italia dalla crisi, né di assegnarle nuovamente il giusto ruolo in Europa. Per questo riteniamo che il dibattito debba prevedere anche nuove fonti di risorse proprie europee, come l'emissione di titoli, sia come integrazione dei meccanismi di intervento in caso di crisi, sia a sostegno della crescita. Vorrei a questo proposito citare un passaggio del Libro bianco del 1985: «L'Europa si trova ad un bivio: andare avanti, con risoluzione e determinazione, o ricadere nella mediocrità. Possiamo decidere di portare a termine l'integrazione delle economie europee oppure, per mancanza della volontà politica necessaria ad affrontare gli enormi problemi che ne derivano, lasciare che l'Europa si sviluppi semplicemente in una zona di libero scambio». In questo In questo senso, il nostro vuole essere un preciso richiamo al senso di responsabilità di tutti ed in primo luogo delle forze di Governo, perché se sceglieremo di non agire rapidamente ed efficacemente e di sottostare al dominio di Paesi economicamente più forti, a partire dalla Germania, non solo l'Italia, ma anche l'Europa si potrebbe ritrovare priva del futuro che le spetta. Signora Presidente, per tutti questi motivi riteniamo positiva la discussione odierna volta a cercare di mettere a punto politiche comuni chiare e sostenibili. Anche attraverso dibattiti politici preliminari, come quello

Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, l'esperienza recente della crisi economica e finanziaria che ha investito l'economia mondiale ha posto all'attenzione dell'Unione europea l'esigenza di realizzare una vera convergenza, sia di bilancio che macroeconomica delle diverse economie nazionali,

volte a rafforzare il Patto di stabilità e di crescita e ad introdurre meccanismi volti a correggere squilibri macroeconomici.

La Commissione affari esteri, in particolare, nel parere che ha reso alla Commissione bilancio, ha rilevato come il complesso di misure in questione implichi, per un efficace governo dell'economia, un'ulteriore cessione di sovranità all'Unione europea. È assolutamente opportuno, dunque, che il Parlamento, come stiamo facendo, si esprima nel merito sui principali temi connessi alla riforma della *governance* economica europea, al fine di conferire un sostegno al Governo, in fase di discussione e di costruzione del rapporto finale della *task force*. Svolgo, quindi, alcune rapide riflessioni sulle principali questioni emerse che dovrebbero trovare uno spazio in sede di definizione e di votazione della risoluzione da parte di questa Assemblea parlamentare. l'analisi della sostenibilità, il rafforzamento della sorveglianza delle politiche di bilancio comporta una maggiore attenzione al debito e, soprattutto, alla sostenibilità fiscale. Tra i parametri di valutazione della sostenibilità di un Paese membro, trovo condivisibile che l'approccio sia ispirato ad una visione di insieme, non per ragioni di convenienza, appartenendo ad un Paese come come l'Italia, con un alto debito in rapporto al PIL, ma per ragioni tecniche. Il concetto di sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e lungo periodo implica un richiamo a fattori ulteriori rispetto al mero debito pubblico, come faceva osservare il senatore Garavaglia nella sua relazione: l'invecchiamento della popolazione, l'andamento delle spese pensionistiche, il livello dell'indebitamento delle famiglie. Quindi, a questo proposito, apprezzabile è stato il contributo del Governo italiano: immagino che si sia trattato di un negoziato difficile, ma ha arricchito il dibattito in sede europea. Su questo punto, la risoluzione dovrebbe dare atto del contributo offerto dal nostro Paese, ribadendo l'opportunità di non limitare l'analisi della sostenibilità all'andamento del deficit e del debito pubblico. Ciò non vuol dire, naturalmente, sottovalutare l'impegno ad una seria riduzione del debito. Occorre anche riconoscere che l'impianto complessivo del Patto di stabilità e crescita ha finora posto un accento prevalente sulla riduzione del deficit e che, fino al 2008, il perseguimento di un obiettivo di riduzione del deficit, in presenza di una crescita nominale del PIL sostenuta, è stata compatibile con la riduzione del rapporto tra debito e PIL. È stata la rapida flessione del PIL, per la congiuntura economica che conosciamo, che ha fatto davvero comprendere il grado di separazione tra obiettivi di riduzione del deficit e del debito. indicare nella risoluzione l'orientamento positivo del Senato ad una visione più ampia della sostenibilità delle finanze pubbliche mi sembra appropriato e non inficia la responsabilità di di ridurre il debito in modo significativo nel medio e nel lungo termine. Quanto alle regole numeriche sul debito, condivido l'opinione negativa sulla proposta della Commissione europea di introdurre una regola numerica sul debito, pari a un ventesimo della differenza tra il rapporto debito/PIL del Paese e il livello del 60 per cento. Il rapporto della *task force*, saggiamente, non contiene alcun riferimento a indicatori numerici. Esso rinvia ad altra sede la definizione di criteri e di metodologia. Ritengo essenziale, però, sottolineare il principio che, nella fissazione di regole numeriche del debito, si tenga conto di un obiettivo di medio termine. D'altro canto, è noto che gli strumenti per agire sulla dinamica del debito sono l'avanzo primario, la crescita nominale e i proventi di eventuali dismissioni del patrimonio pubblico, come è stato largamente osservato anche nel dibattito in Commissione. Prima di stabilire regole numeriche sull'avanzo primario è opportuno, a mio modo di vedere, valutare tutte le ricadute interne in un dialogo stretto con il Governo. Occorre, cioè, valutare la fattibilità politica di vincoli rigidi sull'avanzo primario, soprattutto in relazione al ciclo congiunturale sfavorevole. Connesso a tale chiarimento, ovviamente, è il tema delle regole di evoluzione della spesa. Non credo che il Parlamento disponga ora di tutti gli elementi per comprendere le implicazioni di tale vincolo, prima di aver avviato un confronto approfondito La stessa indeterminatezza contenuta nel rapporto della *task force* suggerisce di rinviare una definizione di dettaglio ad un successivo approfondimento. alle sanzioni e al tema del modello di gestione delle crisi di tipo europeo. Ritengo opportuno che il ruolo delle sanzioni venga in questa fase attenuato e la mediazione raggiunta nel documento della *task force* appare di grande equilibrio. Mi sembra che la gradualità indicata nel documento sia apprezzabile e che ciò debba essere sottolineato nella risoluzione, mentre l'istituzione di un quadro di risoluzione delle crisi, fortemente voluto da Francia e Germania, che richiederebbe una revisione dei Trattati, risulta nella sua problematicità. Nella risoluzione si dovrebbero sostenere le ragioni di preoccupazione di Paesi come l'Italia, che considerano tale percorso non necessario ed incerto. inoltre esprimere una valutazione negativa sull'ipotesi di sospensione del diritto di voto per gli Stati membri. Sulle autorità indipendenti, un aspetto particolarmente enfatizzato negli atti comunitari concerne la necessità, da parte degli Stati europei, della creazione di organismi pubblici in grado di elaborare analisi e previsioni economiche indipendenti. Questo passaggio ci sollecita a riprendere il tema, già affrontato in una prospettiva istituzionale e politica tutta interna al Paese e all'equilibrio dei poteri tra esecutivo e legislativo. Questo passaggio andrebbe assunto ora, in qualche modo per superare quegli ostacoli che fino ad ora hanno impedito la costituzione di un Servizio del bilancio del Parlamento italiano. Ovviamente questa è una problematica che è rivolta al Governo e alle sue competenze. Resta naturalmente - e concludo, signora collegata a questa riflessione il tema della crescita che è intimamente connesso con il piano di riforme strutturali che il Governo e il Parlamento hanno impostato ed avviato in questa legislatura e che devono proseguire, magari con più forza e consapevolezza, sapendo che la dinamica di integrazione dell'economia europea ci costringe ad un percorso virtuoso che può restituire una prospettiva di crescita al nostro Paese, recuperando quei fattori che oggi ci condizionano negativamente, ponendo un argine al debito e favorendo contestualmente quei fattori che aiutino lo sviluppo. Naturalmente sarebbe auspicabile, come è stato anche affermato in molti interventi in Commissione, un'ampia convergenza tra le forze di maggioranza e di opposizione tra le forze di maggioranza e di opposizione su questi temi che riguardano il futuro del Paese, per dare al nostro Governo più forza di negoziare nell'interesse supremo della nostra comunità.

Signora Presidente, ho ascoltato con interesse la relazione del senatore Garavaglia sulla sorveglianza macroeconomica, sulla spesa pubblica, su debito, sanzioni, indicatori di rischio macrofinanziario, come pure sull'inserimento degli immobili sul PIL, che probabilmente avrebbe prevenuto ed evitato la crisi. Spesso però quando si parla di tali questioni, che sono importanti, dimentichiamo il punto di vista dei cittadini, dei risparmiatori, dei contribuenti, che subiscono gli effetti di questa architettura finanziaria. Proprio domani, a poche centinaia di metri dal Senato, in Piazza della Cancelleria, si celebra a Roma l'ottantaseiesima Giornata del risparmio. Secondo una ricerca commissionata dall'ACRI, l'associazione delle casse di risparmio, all'IPSOS, che è un istituto di ricerca - leggo solo i titoli - gli italiani sono preoccupati: uno su quattro si indebita; i consumi crollano; non si toccano sanità, scuola e pensioni; meglio i soldi in tasca, ma l'ideale investimento è quello del mattone. Abbiamo già ceduto pezzi di sovranità all'Europa: pezzi di sovranità che spesso non sono stati utilizzati per gli interessi di questo Paese.

Voglio ricordare che la crisi dei mutui *subprime* non è stata la causa dell'attuale fase recessiva mondiale, ma il sintomo di una grave malattia del sistema economico globale, che è esplosa tramite la finanziarizzazione dell'economia, la creazione del denaro dal nulla, l'inefficacia dei controlli, la collusione tra banche, autorità vigilanti e agenzie di *rating*, le deleghe in bianco che i Governi ed i Parlamenti democraticamente eletti hanno affidato ad oligarchi

In questi anni i Governi hanno lasciato mano libera ai banchieri ed agli oligarchi, perseguendo un teorema secondo il quale il prezzo da pagare alla crescita sregolata

Non sono state redistribuite neppure le briciole. In questi anni abbiamo consentito il saccheggio ambientale e la speculazione sfrenata. La crisi finanziaria ha messo in luce una totale inadeguatezza dei meccanismi di sorveglianza nel prevenire con efficacia l'indisciplina di bilancio, l'esplosione dei debiti sovrani, gli squilibri commerciali e i divari di competitività tra i Paesi membri. Ricordiamo che la Commissione il 29 settembre aveva adottato alcune misure che contenevano una riforma del Patto di stabilità e delle *governance* economiche dei Paesi dell'euro. Quelle disposizioni - poi superate, lo dirò dopo - miravano a rafforzare le procedure di sorveglianza sulle politiche fiscali e prevedevano la riforma del Patto di stabilità e crescita e un'estensione della sorveglianza agli squilibri macroeconomici e strutturali. Un primo elemento di novità riguardava la prevenzione degli squilibri di finanza pubblica. Tutti i Paesi avrebbero dovuto concordare obiettivi di bilancio di medio termine e fino al loro raggiungimento contenere la crescita della spesa pubblica al di sotto della crescita di medio termine del PIL. Era un'innovazione positiva. Accanto alla soglia del deficit del 3 per cento del PIL era introdotto il criterio del debito pubblico che deve convergere al 60 per

Per una volta il compromesso raggiunto potrebbe sfociare in un equilibrio tra l'esigenza di porre sotto controllo i bilanci degli Stati membri e l'obiettivo di non minare la già precaria prospettiva di crescita nell'area dell'euro. Accanto a questo, venivano rafforzati alcuni strumenti di monitoraggio e di controllo delle politiche nazionali di bilancio da parte delle istituzioni europee varati prima dell'estate, nell'ambito degli interventi di sostegno alla Grecia e agli altri Paesi a rischio, sommandosi con i meccanismi europei di prevenzione delle crisi: strumenti che getterebbero le basi per politiche fiscali coordinate tra gli Stati membri, e costituirebbero così il primo mattone per un'Unione non solo monetaria. Giova però ricordare che abbiamo, secondo gli

di 7,1 miliardi al mese: il doppio di quanto era cresciuto negli anni precedenti. Il fatto di aver tolto dal tavolo del negoziato una logica sanzionatoria è un atto di buonsenso soprattutto per il Governo italiano, che riteneva di essere particolarmente penalizzato da criteri automatici di riduzione del debito. per l'Italia la garanzia del rigore fiscale, a cui comunque deve sottoporsi, dovesse avvenire in un contesto di crescita spinta dall'estero, anziché di stagnazione economica. Il Governo è, d'altra parte, certamente alleggerito dall'esser riuscito a far adottare criteri interpretativi del debito che lasciano spazio anche alla considerazione del livello del risparmio privato: quel risparmio a qualche centinaia di metri da qui. La Germania ha ottenuto che il meccanismo utilizzato per il salvataggio della Grecia non sarà prolungato oltre il 2013. Per quella data Berlino vuole una modifica dei Trattati e un nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi che riduca l'eventualità di nuovi interventi pubblici e coinvolga attori privati. Inoltre, ha chiesto l'applicazione di sanzioni politiche molto gravose, come il ritiro del diritto di voto del Paese fuori regola dalle decisioni comuni. In coerenza con tali obiettivi, il meccanismo che è stato proposto dalla Commissione prevedeva che i Paesi il cui debito pubblico superasse il 60 per cento del PIL operassero una riduzione automatica della parte eccedente per un ventesimo l'anno.

*(PD)*. Signora Presidente, lo avevano detto in molti nel corso della grande recessione del 2008-2009 e tutti, poi, lo abbiamo ripetuto, non so quanto convintamente: dopo questa crisi, nulla sarà come prima. La questione di cui ci stiamo occupando, vale a dire sedi, regole, strumenti e obiettivi per il coordinamento delle politiche fiscali ed economiche dell'Unione europea e, in particolare, dell'area dell'euro (perché è di questo che ci stiamo occupando, anche se - me lo lasci dire, signora Presidente - non si direbbe), ci dice quanto quella previsione fosse fondata. previsione fosse fondata. Nel processo di costruzione di una politica economica e di bilancio europea hanno potuto più questi due drammatici anni di crisi, fino allo spettro del fallimento dell'Unione monetaria, che quasi venti anni di auspici circa l'esigenza di associare al mercato unico, prima, e alla moneta unica, dopo, politiche economiche e di bilancio unitariamente definite e robustamente coordinate alla dimensione europea. I Governi nazionali, fino a ieri chiusi ad ogni ipotesi di effettivo coordinamento, oggi stanno, non solo progettando, ma concretamente e rapidamente adottando misure che fino a ieri avevano persino rifiutato di considerare come ipotesi Già si prospettano ulteriori revisioni dei trattati, non per far retrocedere il processo di coordinamento e di armonizzazione delle politiche, ma esattamente per l'opposto, e cioè per accelerarne il passo. Dunque, almeno da questo punto di vista - e, forse, solo da questo punto di vista - sia benvenuta la grande recessione! Le novità che ci si prospettano sono numerose e di enorme portata - me lo lasci dire, signora Presidente - anche se non si direbbe. Vorrei concentrarmi su quella che ritengo la più importante: l'introduzione di un nuovo meccanismo di sorveglianza sui grandi squilibri macroeconomici, ben al di là dell'attenzione fino ad oggi riservata esclusivamente agli andamenti di finanza pubblica (disavanzo e debito) dei singoli Paesi. Non è, colleghi, una decisione da prendere; si tratta di una decisione già presa: d'ora innanzi, la posizione di squilibrio eccessivo di uno Stato membro su dati macroeconomici, come la bilancia dei pagamenti correnti e commerciali o le dimensioni del settore immobiliare rispetto al prodotto,

La Commissione e la *task force* del Consiglio europeo partono da una comune consapevolezza: il Patto di stabilità e crescita non si è rivelato sufficiente né a garantire la stabilità né a favorire la crescita.

Su alcune di queste questioni fondamentali decideranno le istituzioni comunitarie, a partire dal Consiglio europeo di domani e dopodomani. Sappiamo già, tuttavia, qual è il novero degli indicatori tra il rapporto tra saldo delle partite correnti e prodotto. Cosa c'è dietro questa scelta? Se un Paese domanda stabilmente più di quello che produce determina nel contesto dell'Unione monetaria squilibri capaci di contagiare l'intera area monetaria di cui fa parte. L'Italia su questo punto non sta affatto bene.

sette punti in meno nel corso di questi 15 anni segnalano chiaramente uno squilibrio strutturale della nostra economia. È molto grave.

del risparmio e della ricchezza patrimoniale. Un criterio, quello del debito privato, assolutamente sacrosanto per valutare la stabilità di un sistema; ma non inganniamo la gente, i cittadini italiani. Questo criterio - che va introdotto - è parallelo, non incide, non modifica e non depotenzia il criterio sul debito pubblico che, anzi, verrà potenziato in termini di esercizio dell'attività di sorveglianza.

la nostra è stagnante da 15 anni e questo causa una scarsissima capacità di attrarre investimenti esteri ed una progressiva perdita di capacità competitiva.

del sistema in passato, sono state il debito pubblico e le svalutazioni, non la bolla immobiliare, che da noi non ha avuto un'esplosione analoga a quella che si è registrata Come si vede, dunque, convivono nel nostro sistema economico fattori di forza e di equilibrio con indicatori drammatici di uno squilibrio molto grave e molto serio. È dannoso e diseducativo raccontare agli italiani che è possibile, nelle decisioni europee, deprimere il peso degli indicatori che ci vedono in posizione di squilibrio, esaltando invece quelli che segnalano equilibrio.

fuoco! Non abbiamo dunque alternative. Dobbiamo fare subito riforme coerenti dei mercati dei fattori: mercato del lavoro, infrastrutture e servizi in rete, energia, educazione, formazione e ricerca, pubblica amministrazione e giustizia, apertura dei mercati chiusi e liberalizzazioni. Sono riforme che, anche se fatte subito e bene, tarderanno a manifestare i loro effetti positivi in termini di innalzamento delle capacità competitive e della qualità sociale del nostro sistema, ma bisogna agire subito: ce lo dice l'esperienza che abbiamo fatto in questi lunghi anni. Il documento della *task force* del Consiglio indica due fattori di rischio per la sostenibilità della finanza pubblica per i quali la posizione dell'Italia è relativamente migliore. l'invecchiamento della popolazione, per l'effetto che provoca sui sistemi pensionistici quando siano - e purtroppo lo sono diffusamente - troppo generosi verso i *baby boomer*, cioè verso la mia generazione. luogo, il salvataggio pubblico di istituti bancari per l'aumento del debito concentrato nel tempo che esso ha determinato. Ebbene, se oggi il nostro Paese è in una posizione migliore rispetto a questi due fattori di rischio,

dunque è chiara, e dovremmo finalmente deciderci a tirarla tutti assieme: fare le riforme paga; non farle si paga, e si paga molto salato. Lavoro, giustizia, professioni, pubblica amministrazione, energia, infrastrutture materiali e immateriali, mercato del lavoro:

usare il vincolo europeo per forzare il Paese ad accettare cambiamenti troppo a lungo rifiutati. Abbiamo un primo appuntamento: entro il 12 novembre il Governo dovrà presentare alla Commissione la bozza del Piano nazionale delle riforme:

Quali riforme, in quale ordine di priorità, per quali ben definiti e verificabili obiettivi, anche espressi in termini numerici, quantitativi? Chiediamo al Governo - lo faremo anche con la nostra proposta di risoluzione - di impegnarsi adesso, qui, di fronte al Senato, di avviare, partendo dalla discussione su questa bozza di Piano nazionale delle riforme da presentare entro il 12 novembre, un confronto che coinvolga l'intero Paese, facendo uscire la politica italiana

che ci si apre dinanzi è dunque una fase difficilissima e irta di difficoltà, ma anche di enormi potenzialità per la soluzione dei problemi strutturali del Paese, compreso quello della organica incapacità di mettere sotto controllo la crescita della spesa corrente primaria (negli ultimi 10 anni, più 4,6 per cento all'anno, ogni anno rispetto all'anno precedente). Non è questione che si risolve con provvedimenti di emergenza e con misure tampone. Ci vogliono regole rigide di evoluzione della spesa in proiezione pluriennale. Il nostro Gruppo aveva lungamente insistito senza successo per prevedere specifiche regole di evoluzione della spesa nella legge di contabilità nazionale che abbiamo votato nel 2009. Allora, il Governo si era opposto, ma non è stata una buona scelta. Tra pochi giorni lo stesso Governo, lo stesso Ministro verranno a chiederci di modificare proprio in questo senso la legge n. Non è solo questione di rivendicare una primogenitura (sia ben chiaro: noi avevamo visto giusto, il Governo aveva visto sbagliato); è soprattutto questione di tempestività delle scelte di riforma. Ogni ritardo viene pagato dal Paese, esattamente come accadrà, se ancora permarrà a lungo lo stallo sulla costituzione di una istituzione-organismo indipendente di valutazione e analisi dei conti pubblici. Trasparenza ed attendibilità dei conti pubblici, come ha dimostrato anche ai ciechi la tragedia della Grecia, costituiscono un fondamentale bene pubblico. Ora, sia la Commissione sia la *task force* del Consiglio raccomandano la costituzione di questi organismi a dimensione nazionale, scrivendo nei loro documenti che ciò è essenziale per «assicurare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche». Cosa deve ancora accadere, colleghi della maggioranza, per convincerci a fare subito quel Servizio del bilancio del Parlamento italiano sul modello del CBO statunitense che quest'Assemblea ha più volte mostrato, col voto e non con le parole, di considerare indispensabile? Subito vuol dire subito. Lo raccomanda l'Europa. Lo pretende lo stato di clamorosa ignoranza in cui tutti noi versiamo, io per primo, in tema di dati indispensabili per l'attuazione della legge sul federalismo fiscale. Infine, la richiesta al Governo di impegnarsi in Europa ed in altre istituzioni del governo globale perché i frutti di questo sforzo di superamento degli squilibri globali, che minacciano stabilità e qualità dello sviluppo, possano dar luogo ad inedite forme di gestione europea del debito pubblico e ad investimenti europei sulle infrastrutture, materiali e immateriali, sostenute da emissioni di titoli di debito pubblico che godano dell'accresciuto merito di credito dell'area dell'euro. Il ragionamento è semplice: se tutti i Paesi se tutti i cittadini di tutti i Paesi europei sopporteranno il peso -perché saranno pesanti, colleghi, molto pesanti delle politiche di superamento degli squilibri e se queste politiche avranno successo, il merito di credito del sistema euro nel suo complesso migliorerà. È la circostanza migliore per realizzare l'ipotesi lungimirante del grande presidente Delors: *eurobond* per finanziare investimenti in infrastrutture, materiali e immateriali, di rilievo europeo. Allo stesso modo, la definizione di regole comuni per la nuova *governance* economica europea può favorire, ed anzi ne costituisce il necessario presupposto, soluzioni per la gestione comune del debito pubblico.

un fondo che potrebbe finanziarsi anche con quel prelievo sulle transazioni finanziarie a breve che, adottato a dimensione internazionale, vince le obiezioni circa la sua praticabilità nella dimensione nazionale.

Non vogliamo accettare il commissariamento del nostro Paese da parte di un unico Ministro che partecipa alle decisioni europee e che ha commissariato anche il resto del Governo. Il Governo tecnico c'è già, non bisogna farlo. C'è già. *(Applausi dal Gruppo PD).* Ma le scelte che andremo a fare domani in Europa riguardano il sistema-Paese e influenzeranno il futuro del nostro Paese per i prossimi vent'anni. Ne vogliamo parlare qui, perché la nostra è una forma di governo parlamentare. Finché è così, questa è la sede nella quale esercitare la funzione di indirizzo nei confronti delle scelte del Governo. *(Applausi

perché la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di associare l'esame di una serie di documenti così importanti a quello di una mozione parlamentare,

si lamentino, giustamente, di non affrontare le questioni fondamentali della vita nazionale e quelle che impattano sull'economia e sulle questioni sociali, quando, obiettivamente, il dibattito che stiamo svolgendo stiamo svolgendo è, appunto, parte molto rilevante di ciò che preoccupa i cittadini, le imprese, le famiglie e il sistema produttivo nazionale. Vi è un argomento che potrebbe tenere insieme

che spesso ha aiutato l'Italia a tagliare traguardi importanti, e il commissariamento, inteso come commissariamento europeo. Verrò tra un attimo al tema sollevato in chiusura dal collega Morando a proposito di ciò di cui - sottosegretario Casero - ci si occupa nel Parlamento, e della misura con la quale il Governo, guidato per la politica economica dal ministro Tremonti, porta davanti al Parlamento non le decisioni che contano, ma una collana di eventi e di provvedimenti, che di volta in volta trattano una piccola parte dell'insieme e non ci permettono mai di affrontare l'insieme. parliamo di stabilità e di crescita. Il tema della crescita, si ricordava poc'anzi, il Parlamento lo dovrebbe affrontare di qui a due settimane,

nell'orizzonte del patto per la crescita al 2020. Cioè, si affronta la crisi economica e

Dove si incontrano allora queste due problematiche, cioè gli argomenti all'ordine del giorno del Senato e la mozione che, assieme agli altri colleghi, avevamo presentato, e che la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto di associare? Perché la nostra mozione è tutta interamente incentrata sulla problematica della crescita, naturalmente possono essere discusse, che possono essere parzialmente o interamente condivise dal Senato, ma che comunque toccano il problema numero uno. Qui apro un unico fronte

Ci fu detto all'inizio della legislatura che la politica economica era stata, tutto sommato, inquadrata attraverso un provvedimento che il Consiglio dei ministri aveva approvato in nove minuti e che, da quel momento, la legge finanziaria sarebbe stata una formalità. Bene, lo ricordava adesso il collega Morando, la legge di contabilità e finanza pubblica approvata nel dicembre dello scorso anno è già da buttare. Ma il punto è un altro: oggi il Governo (alcuni Ministri, per la verità) ha annunciato che dopo che abbiamo approvato l'ex DPEF

prima della fine dell'anno. Il Governo dovrà affrontare gli indirizzi del Parlamento sulle politiche per la crescita al 2020 richieste dagli appuntamenti europei che ho appena ricordato, ma annuncia anche la presentazione di un cosiddetto decreto milleproroghe. la politica economica e quella di bilancio si fanno con decreti-legge. Sappiamo che il milleproroghe, correggetemi se sbaglio, lo scorso anno è valso circa 9 miliardi di euro: quindi, una delle parti principali della manovra annuale è stata fatta attraverso il decreto milleproroghe. Alla fine di quest'anno ci aspettiamo un preannunciato decreto-crescita, nel quale alcuni Ministri intendono inserire risorse (esempio quelle per la cultura, magari quelle per l'università, che sono carenti e non vengono inserite bizzarramente laddove dovrebbero, cioè nella manovra che oggi si chiama legge di stabilità); in più, arriverà il milleproroghe, che diventa quel treno al quale ciascuno aggiungerà i vagoni di interesse per tappare altri buchi e fronteggiare altre evenienze, sempre di natura strutturale e certamente non marginale. Dunque, siamo dinanzi ad un quadro drammatico, signora Presidente, che è il seguente: l'Europa si interroga su come l'Italia sia in grado di onorare i propri impegni in materia di politica economica e di stabilità della nostra macroeconomia e dei suoi orizzonti, e noi cosa facciamo? Qual è la risposta dell'Italia? Qual è la riposta del nostro Paese in ordine alle priorità per la crescita,

se ce ne saranno - come mi auguro - le condizioni, un indirizzo per realizzare la crescita economica, e non soltanto la presa d'atto presa d'atto (come hanno ricordato tutti i colleghi che sono intervenuti della maggioranza e dell'opposizione), cui ci troveremmo al termine di questo dibattito di dover provvedere sulle regole europee che impattano su di noi. Abbiamo anche osservato come la semplice applicazione di alcune delle sanzioni ipotizzate in caso di inadempienza delle norme che ci accingiamo ad adottare in sede europea avrebbe per il nostro Paese un impatto gigantesco. Ed allora, dovremmo spiegarci meglio, e la domanda che io rivolgo al Governo é

alla riunione dei suoi colleghi per capire come vada a finire una vicenda che l'ultimo vertice europeo ha consegnato ad una decisione insoddisfacente (con il compromesso tra il Governo tedesco e quello francese), cominciare da questo dibattito per dire, auspicabilmente maggioranza e opposizioni, che l'Italia deve imboccare la strada della crescita economica, se vuole immaginare di centrare gli obiettivi, virtuosi virtuosi o per costrizione, della stabilità economico-finanziaria. Questo è il tema, signora Presidente, che noi intendiamo porre nel documento che abbiamo presentato, ricordando che l'Italia si presenta a questo appuntamento con una crescita della spesa, al netto degli interessi, inquietante; che l'Italia si trova con una crescita della spesa regionale inquietante Garavaglia, che la vera messa in discussione del radioso orizzonte - come viene presentato da alcuni - del federalismo risiede esattamente in questo. Noi avremo cioè un federalismo con restrizioni, non un federalismo bengodi che dà al Nord la possibilità di liberare le proprie energie e al Sud nessun aggravio rispetto alle condizioni drammatiche in cui si trova. Un federalismo immaginato con questo quadro di restrizioni che non può - come sta già accadendo con la manovra di quest'anno - che andare a toccare pesantemente i trasferimenti alle Regioni e agli enti locali, e sarà ben diverso da quelle che, in particolare la Lega, ma anche altre forze politiche in quest'Aula, hanno inteso presentare ai loro elettori per i prossimi anni. In ciò scorgo, collega Morando, uno degli elementi cruciali che potrebbero portare alla fine della legislatura.

ma appropriatamente al 2020, dovremmo discutere di quelle misure strutturali che ci consentano di recuperare competitività, così come produttività e vigore e dinamismo dal punto di vista economico. E quale riforma più importante di quella dell'università e della ricerca dovrebbe consentire all'Italia, da qui ad un decennio, di rimettersi in carreggiata in termini di crescita? In questo passaggio è contenuta la contraddizione più lampante, signor rappresentante del Governo, con un Parlamento che approva una riforma (che non tutti hanno condiviso: noi sì), ma sapendo bene che si sarebbe poi arrivati rapidamente al momento della verità in cui si sarebbe appurato se le risorse ci sono o non ci sono. Nel momento in cui la riforma viene rimandata, messa nel *freezer* perché le risorse non ci sono, emerge la contraddizione di un Paese che è catturato, imprigionato tra le esigenze della stabilità e i ritardi incapacità di saper scegliere, di fare gli investimenti in quei comparti che servono a far ripartire la crescita, non solo e non tanto nel breve ma nel medio e lungo termine, quale certamente la riforma dell'università. Qui vien fuori la contraddizione di un Ministero che fa tagli lineari, alla pari, in tutti i comparti, anziché scegliere dove si deve colpire. Indiscutibilmente, ci sono aree nelle quali dolorosi tagli sono non solo indispensabili, ma possibili e delle aree in cui sono impossibili, assurdi, controproducenti come quello che ho appena citato. Signora Presidente, parliamo di un Paese, il nostro, che non ha la gente in piazza sulla riforma delle pensioni, che ha già fatto ed in misura più coraggiosa di quella del Governo francese. Questo va detto ad onore dei Governi precedenti e del senso di responsabilità delle forze sociali,

anni. Dobbiamo creare le condizioni per il ritorno alla crescita, altrimenti, di cattura in cattura, saremo soltanto catturati dentro l'automaticità delle sanzioni

tanto cruciale per tutti i comparti produttivi del nostro Paese. Inoltre, potrei citare l'Esercito europeo, in un momento nel quale in tutta Europa i grandi Paesi, a partire da quelli che hanno l'arma nucleare (Francia e Regno Unito), tagliano drammaticamente il bilancio della difesa senza porsi il problema che forse è arrivato il momento, più che di tagliare i bilanci nazionali, di stabilire una procedura che porti l'Europa ad avere un Esercito europeo credibile a livello internazionale,

alla luce di queste considerazioni, si inserisce bene nel nostro dibattito, perché chiede che il Governo e il Parlamento concentrino l'azione nella seconda metà della legislatura su riforme e provvedimenti mirati alla promozione della crescita economica impegna il Governo a promuovere le iniziative che concorreranno a formare l'agenda per la crescita e il programma nazionale di riforma per la strategia europea «per l'occupazione ed una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» nel decennio 2010-2020. La nostra mozione introduce molte proposte (che semplicemente elenco senza descrivere), a partire dai tagli dei costi della politica.

ad assumersi una parte di ridimensionamento dei propri costi nel momento stesso in cui lo chiede alla società produttiva del nostro Paese. Indiscutibilmente la *spending review* deve essere fatta sulla base di parametri mirati. al taglio dei margini di spreco e di inefficienza nella sanità, che ci sono ancora; al disboscamento (questa è la prima parte della mozione, quella che riguarda il taglio della spesa) dei finanziamenti pubblici improduttivi alle imprese, oggi distribuiti a pioggia; all'accorpamento delle Province e alla ridefinizione dei compiti degli enti territoriali; ad un federalismo competitivo, che sia cioè in grado anche di consentire agli utenti di scegliere i servizi migliori e comporti premi per le prestazioni più efficaci. Il secondo capitolo concerne il miglioramento della competitività del sistema. Nel nostro testo si citano tre documenti che possiamo definire europei:

sulle liberalizzazioni e il rapporto della Banca d'Italia sul Mezzogiorno. A nostro avviso, i tre temi sul Mezzogiorno, sulle liberalizzazioni e sul mercato interno, con riferimento a documenti di istituzioni nazionali, al massimo livello di autorevolezza, od europee possono essere una chiave d'intervento forte e convincente. Nella mozione si parla poi della questione giovanile, riferita all'accrescimento di opportunità, soprattutto con riguardo alle professioni, giustizia, che fa parte delle politiche per la competitività e non solo della rissa quotidiana per affrontare di volta in volta un lodo

tagli della spesa pubblica, a proposte per i comparti manifatturieri, per il *made in Italy* in particolare, per la scuola, l'educazione, la conoscenza, la ricerca, l'agenda del digitale, il programma per le piccole, medie e grandi infrastrutture, l'economia verde infine per il contrasto della corruzione e la crescita della produttività, considerati come fattori decisivi per il recupero della competitività. In conclusione si fa riferimento alla questione demografica, alla famiglia e al ruolo della società nella ripresa della crescita economica del nostro Paese. In sintesi, signora Presidente, onorevole collega relatore, signor rappresentante del Governo, cogliere l'occasione di questo dibattito nel quale ci troviamo con il fucile puntato delle nuove regole europee sulla stabilità della nostra finanza pubblica per farne anche un'occasione per fornire i primi indirizzi per la crescita. C'è la possibilità che vi sia una condivisione tra maggioranza e opposizione? Me lo auguro, come mi auguro ci siano altre proposte che, in sintonia o anche in parziale dissenso da quelle contenute in questa mozione, ci permettano di fare del dibattito odierno un dibattito costruttivo ed utile per il Paese.

Francamente ciò che dirò sembrerà in entrambi i casi fuori tema, pur essendo io profondamente convinto che fuori tema

collega Rutelli e che tutte le persone ragionevoli e di buon senso in tutta Europa ma anche nel resto del mondo possono capire), non si va da nessuna parte con dirompenti squilibri finanziari, con dilaganti deficit e debiti pubblici.

Il tema é: come si può raggiungere l'equilibrio finanziario in termini strutturali? E allora viene in ballo il problema della crescita economica. Se è vero che senza equilibrio finanziario non c'è crescita economica, ma c'è pia illusione, è altrettanto vera e sullo stesso piano altrettanto vera e sullo stesso piano l'affermazione che, senza crescita economica, non c'è equilibrio finanziario. Signori banchieri d'Europa, è nel vostro interesse che, ovviamente, guardiate di più all'equilibrio finanziario e all'andamento dei debiti pubblici perché, in gran parte, quei debiti sono nell'attivo dei vostri patrimoni. Quindi, ciò è giusto, ma sappiate che, se chiedete e pretendete dall'Europa soltanto l'equilibrio dello strozzino, anche i vostri bilanci salteranno, perché senza crescita non c'è equilibrio finanziario. Questo è il tema che l'Europa si deve porre in termini di *governance*. Allora, signora Presidente, una semplice constatazione. Qual è l'attuale *governance* europea? Quale è l'attuale politica economica europea? Da un lato, la Banca centrale europea è bloccata dal suo statuto. Non è certo colpa del presidente Trichet, ma di quanto è scritto nello statuto, che ha visto assegnare alla Banca centrale europea esclusivamente l'obiettivo del controllo dell'inflazione sotto o, comunque, attorno al due per cento. Punto! Questo prevede lo statuto della BCE. Ed è uno statuto talmente stupido da non capire un fatto elementare, che da 70 anni è scritto su tutti i testi di economia: l'inflazione si può controllare, ma ciò che va considerato è a quale costo questa si controlla in termini di crescita economica. Io sono in grado di portare l'inflazione a zero, con una crescita a meno cinque per tre anni consecutivi; anzi, di portarvi sotto zero, alla deflazione. Ma questo neanche gli studenti del primo anno di economia si permettono di dirlo! Purtroppo, però, i soloni europei guardano con un occhio solo. Faccio l'esempio più banale. Se quello statuto che impone alla BCE di controllare l'inflazione,

trascurare il fatto che il renminbi cinese è agganciato politicamente al dollaro americano. Quindi, noi regaliamo alla Cina, oltre al suo *dumping* sociale, questo 30-40 per cento, che non costa nulla a nessuno, salvo a noi europei. nel momento in cui la BCE guida la macchina della politica monetaria con un occhio solo, essa controlla l'inflazione e determina, in queste condizioni, due punti in meno di crescita media in tutti i Paesi europei.

che, di fatto, si è spostato in Cina e, in parte, negli Stati Uniti; ma non per una sana competizione di mercato aperto, non per una globalizzazione con regole condivise, ma per una stortura, per una distorsione: quella cioè di aver consentito ad un grande Paese come la Cina di entrare nel commercio (cosa giusta e santa), senza ribadire, in contropartita, che se si entra nel libero scambio delle merci bisogna entrare anche nel libero scambio delle monete. si bloccano i prezzi, è ovvio che si determinano squilibri nelle quantità. È questa ragione perversa che toglie all'Europa il 2 per cento all'anno di crescita! stiamo a guardare, come gli entomologi guardano le ali delle farfalle, se la ripresa è del più 0,6 o del più 0,7

le due grandi economie manifatturiere europee, Germania e Italia, hanno avuto immediatamente il rimbalzo nelle esportazioni. Ma di che stiamo parlando, cari colleghi? E questa è la linea della politica monetaria della BCE. Non è un fatto personale con il presidente Trichet, è un fatto collettivo, politico: bisogna cambiare lo statuto della BCE! all'altra gamba, la politica di bilancio (quella che certi colleghi anglofoni definiscono *fiscal policy*: in italiano si direbbe politica fiscale, ma detto in italiano sembrerebbe la politica delle tasse, mentre in inglese è la politica dell'intero bilancio: spesa, entrate, saldi e quant'altro) affidata a Maastricht 1. Quel sacrosanto patto, necessario per fare l'euro, l'unificazione monetaria, assolutamente necessario e sacrosanto in quel momento, è una regola oggi ridicola.

che può stare fuori casa fino a tardi, che può anche andare in discoteca fino alle tre della notte, però deve bere poco, essere in grado di guidare l'automobile, non rincitrullirsi con le droghe.

E chi è virtuoso e crea un avanzo di parte corrente può fare investimenti pubblici, infrastrutture, ricerca, innovazione. Magari con un rapporto saggio, di uno a uno: se hai l'uno per cento di avanzo corrente puoi fare un 2 per cento di investimenti. E allora in parte gli investimenti possono e debbono essere a deficit. Perché una normale famiglia che deve comperare una casa, è ovvio, per il 70 per cento accende il mutuo. È giusto che si indebiti, ma per la semplice ragione che l'utilità, l'uso di quel bene, è spalmato nei venti-trent'anni futuri e viene consegnato alla generazione dei figli. Le infrastrutture, la ricerca, le innovazioni, vanno viste con un orizzonte temporale di lungo periodo. Non è possibile pretendere che l'Alta velocità ottenga un finanziamento nell'arco di due o tre anni o che opere pubbliche importanti ottengano l'equilibrio finanziario in pochissimo tempo. Perché? Perché il risultato perverso è quello che abbiamo ottenuto, mantenendo Maastricht al tre per cento con l'obiettivo di stare attorno al 60 cento nel rapporto debito-PIL. Ricordo, signora Presidente, che questi numeretti in quel momento vennero fuori come un gioco del pallottoliere. Forse i colleghi lo sanno, forse qualcuno non i nostri *guru* delle burocrazie autoreferenti europee dissero: siccome l'Europa nei prossimi trent'anni avrà un'inflazione del 2 per cento, perché la controlla la BCE, e una crescita media annua del 3

Ridicolo! Perché? Perché l'effetto sulla crescita economica non è determinato dal deficit. È vero che se il deficit è dilagante, la crescita implode, ma non è il deficit che fa la crescita. Ciò che fa la crescita è il livello della spesa pubblica, la sua composizione, la sua ripartizione. Nella spesa corrente, fatemi aggiungere, nel nostro Paese esistono 60-70 miliardi, su voci specifiche che ho più volte denunciato in quest'Aula, di ruberie, di furti, di aree grigie, tra economia, criminalità e politica. Di questo dobbiamo parlare. E allora, nuovo statuto della BCE e nuovo Patto di Maastricht. Questa è la nuova Europa che può determinare, e autodeterminare, le proprie condizioni di crescita economica, altrimenti rimarrà l'Europa asfittica, impotente nel consesso internazionale, che accetta supina un finto G20 che ogni volta che si riunisce decide un centimetro di strada, quando il percorso è di 100 chilometri.

primi. Allora, questa è la conclusione. Di cosa stiamo parlando? Della nuova *governance* europea, cioè di quel pacco di carta straccia piena di burocratese che ci vengono a contrabbandare come il nuovo Patto?

flessibili. Chi mi conosce sa che per trent'anni ho sostenuto l'idea che l'Italia fosse un Paese molto solido, perché a fronte di un debito pubblico aveva un enorme risparmio privato. E ciò che conta in un'economia è il risparmio netto nazionale, è ovviamente la somma dei due settori. Quando avevamo deficit al 10 risparmio negativo pubblico all'8-9 per cento, avevamo famiglie e imprese italiane che producevano un risparmio del 16 per cento! Mai avvenuto nei grandi Stati Uniti d'America; mai! Quindi, è ovvio che quell'elemento del risparmio privato, affiancato al risparmio pubblico negativo, al debito, debba essere valutato. Ma questo significa semplicemente quel che sappiamo da tanti decenni, cioè che gli italiani sono un popolo saggio, mediamente ricco, che sa risparmiare, che sa prendere le decisioni nella propria famiglia e nella propria impresa in modo

a parità di deficit, spostare le risorse significa o consolidare e potenziare, o minare e sgretolare le basi della crescita economica di un sistema,

sono decine e decine di miliardi di euro, dai quali potrebbero derivare decine e decine di miliardi di entrate fiscali fisiologiche, non vessatorie, ma dovute alla crescita e alla prosperità e, quindi, anche al riequilibrio della finanza pubblica. È chiaro che tutto questo presuppone gli Stati Uniti d'Europa politici: non sono chiacchiere da tecnocrati, ma si presuppone una guida politica. So che tutti i colleghi hanno una formazione culturale ben più profonda della mia, ma chiedo (se si potesse farei un sondaggio, anche se siamo pochi) quanti di noi ricordano il nome del Presidente del Consiglio dell'Unione europea o del Ministro degli esteri dell'Unione europea: vagamente si sa che la seconda è una donna e il primo è un uomo. Ma soprattutto, ammesso che ne ricordiamo i nomi,

con singoli interessi, equilibri interni, assi particolari: Est-Ovest, Centro-Sud, Germania-Francia. Si spacca l'asse franco-tedesco e allora c'è un altro asse e si fa la grande Bavaria o altre cose. L'Europa ha urgenza di essere Stati Uniti d'Europa. Capisco i sorrisetti di molti che ritengono questa una pura illusione utopica.

come posso dire? - privilegi o posizioni di casta. Un'ultima osservazione: ho letto attentamente la mozione del collega Rutelli e ne condivido tutti i titoli,

Chiudo, signora Presidente, sul secondo passaggio che lega questo dibattito all'altro: la *governance* europea e la politica economica italiana. È arrivata alla Camera una legge finanziaria tabellare.

è se sia consentito fare proposte di politica economica concrete per le famiglie, per le imprese, per gli investimenti pubblici, per le forze di polizia, per le forze di difesa e sicurezza, per l'università, per la ricerca: questo è possibile, a condizione che ciascuna di queste

dove tagliare le risorse per spostarle e coprire queste esigenze di crescita, di sviluppo e di maggiore giustizia sociale. Infatti, parlare di famiglia vuol dire parlare del nocciolo duro e vero del nostro Paese,

*(PdL)*. Signora Presidente, senatrici e senatori, il periodo dal 2008 ad oggi ha visto in progressione la crisi immobiliare negli Stati Uniti, la crisi bancaria mondiale, il crollo dei consumi, l'aumento della disoccupazione e automaticamente il passaggio dal sistema del privato al pubblico con il trasferimento dei debiti agli Stati. Il trasferimentodei debiti agli Stati è avvenuto con l'esplosione del debito pubblico, in parte per sostenere il sistema bancario o delle imprese e, in parte, quindi, per dare liquidità. Questo ha generato la crisi degli Stati. Il passaggio della crisi è stato dal privato agli Stati. La Grecia è stata in Europa l'esempio più estremo e ha fatto prendere consapevolezza della debolezza dell'Unione europea e, in particolare, dell'area euro. Questi fatti hanno reso evidente che unione monetaria senza unione economica non funziona, che unione economica a questo punto significa avere una *governance* in grado di decidere, avere uno stesso linguaggio di lettura e confronto dei dati (cosa che non c'è in Europa in questo momento), avere dei percorsi decisionali nazionali temporalmente coordinati tra i vari Paesi dell'Unione europea. Da ciò nascono positivamente i documenti e la prima intesa che sia in Commissione che nella*task force* costituita prevedono il semestre di bilancio europeo che dovrebbe portarci ad evidenziare le nostre valutazioni per l'anno successivo nel mese di aprile, al momento della

Si pone per l'Europa ciò che il Parlamento italiano si è posto con la legge di contabilità n. 196 del 2009 e più ancora con la riforma federale.

sappiamo bene che abbiamo realtà dove non riescono a ricostruire i conti della sanità e automaticamente il bilancio regionale), enti locali con bilanci in dissesto e continue emergenze che si riversano a livello centrale. Allo stesso modo, l'Europa e, in particolare, i Paesi dell'area euro sono obbligate dai fatti ad avere economie integrate. Questo stato di crisi, come è già stato detto peraltro sia dal collega Morando che dal senatore Baldassari, determina automaticamente l'obbligo, e non la scelta, di un nuovo modello d'Europa,

a tutto il Paese, ma se un Paese europeo va in *default* fa danni a tutta l'Europa. Non è più possibile ragionare per compartimenti stagni,

burocrazia nei vari Paesi dell'Unione europea. La riforma delle pensioni in Francia non è solo un problema francese che possiamo guardare in televisione dicendo: anche in Francia hanno dei problemi; anche Sarkozy ha le rivolte. La soluzione della questione pensioni francese è un problema anche nostro. ricordare che qualche mese or sono, a causa della crisi greca, in una tumultuosa notte di trattative sulle misure d'intervento, l'euro rischiò di saltare.

se vogliamo mantenere la moneta unica, dobbiamo avere regole uniche, non velleitarie, che possano essere rispettate e cogestite. Per questo è importante che, accanto alle regole, ci sia il controllo del loro rispetto e una *governance* in grado di intervenire tempestivamente.

unica in Europa, di un modello di *governance* che permetta di assumere decisioni politiche tempestive. Noi partecipiamo a questa fase europea, mentre

Molti sono i temi connessi a questo argomento, ma vorrei qui soffermarmi sui temi dell'efficienza del lavoro e sulla competitività delle imprese.

Viene quindi immediato pensare alla riforma del federalismo ed al merito della Lega di aver combattuto per questo e dei cittadini che ci sostengono sempre più numerosi ed in tutto il Paese. Un altro esempio significativo su questo tema, come sistema industriale, sistema industriale, è la Volkswagen. Un esempio virtuoso di accordi sindacali e territoriali, di concorrenza interna tra gli stabilimenti in senso mondiale, specialmente per le scelte che sono state avanzate, sicuramente anche molto pragmatiche con le parti sociali. Vorrei, ad esempio, ricordare le politiche di riduzione del salario, con i contratti di riduzione di salario, la variazione dell'orario di lavoro, le assunzioni differenziate, vedi l'accordo cosiddetto 5000-5000. Non possiamo purtroppo fare le stesse considerazioni se guardiamo i casi locali, iniziando dal rapporto FIAT-sindacati. della proposta della Lega di legare le retribuzioni al costo della vita, che in Italia varia in maniera sostanziale dal Nord al Sud, anche perché i cittadini vogliono cose semplici ed immediate e non certamente sentir parlare solo dei massimi sistemi.

L'idea nasce da un dato di fatto incontrovertibile: l'Italia dal punto di vista economico è un Paese spaccato, con un Centro Nord in cui esiste una disoccupazione bassa e un costo della vita alto e un Sud in cui, al contrario, si ha una disoccupazione a livelli *record* e un costo della vita sensibilmente minore rispetto al resto d'Italia. La proposta è sensata per varie ragioni. Il salario, infatti, non è un'entità astratta, un numero o un concetto matematico puro. In sostanza, il valore numerico in sé è irrilevante (e ce ne siamo anche accorti negli ultimi anni quando, dopo l'adozione dell'euro, gli stipendi, pur rimanendo formalmente identici, hanno perso gran parte del loro potere di acquisto). Su questa base risulta incomprensibile l'assoluta contrarietà che la proposta ha suscitato nei sindacati e nell'opposizione di sinistra che almeno, stando alle dichiarazioni di intenzioni, ha sempre mirato a garantire ai lavoratori il soddisfacimento dei propri bisogni specifici.

che per ridurre questa dualità si dovrebbe puntare all'aumento del numero di occupati piuttosto che all'aumento del salario di chi un lavoro già ce l'ha. Calmierare le retribuzioni su base regionale risulterebbe positivo: i lavoratori del Nord infatti potrebbero godere di una maggiorazione sulle loro buste paga, che permetterebbe loro di garantirsi consumi più adeguati alle proprie esigenze (tonificando in tal modo con un aumento della domanda anche la congiuntura economica), mentre al Sud il minore costo del lavoro consentirebbe di aumentare il numero complessivo degli occupati (in quanto in un sistema ormai globalizzato i posti di lavoro tendono a spostarsi in zone dove il costo è più basso). Criticare le proposte di chi governa, anche quando sono dettate dal semplice buon senso, è una prassi che in Italia sembra quasi essere un obbligo per chi è all'opposizione; tuttavia la difesa aprioristica dello "*status quo*" e la paura di ogni cambiamento, che contraddistinguono i sindacati rischiano di rivelarsi scelte molto dannose. Esistono forti differenze di *status* nel nostro mercato del lavoro, dove a soggetti che godono di ampie garanzie, in certi casi anche eccessive alla luce delle crescenti difficoltà economiche e di cui a volte si abusa, si contrappongono soggetti quali i precari, i lavoratori a tempo determinato e a progetto o gli occupati in piccole imprese, che sono privi di qualunque tutela. Siamo anche intervenuti su questo tema con misure *ad hoc* che hanno dato significativi risultati, ma ovviamente non sufficienti. Quello di cui sto parlando è un sistema strutturale di risposta globale e complessiva. Nonostante questo, le forze della sinistra si oppongono strenuamente a ogni cambiamento che tenda a limitare le garanzie acquisite da alcuni al fine di concederne in parte a chi ne è sprovvisto. In questo paradosso finiscono per assumere un ruolo conservatore, nel senso più letterale e negativo del termine. Ci auguriamo, quindi, che questa modalità del mondo del lavoro e dell'occupazione, che è stata impiegata e attuata anche positivamente con gli esempi che prima ho citato a livello di Paese o di gruppi industriali, possa finalmente trovare

Signora Presidente, possiamo dire che da domani cambia la musica, cioè che sotto la pressione della grande crisi globale cambia la musica: cambia radicalmente il rapporto tra le politiche nazionali e quelle europee, con uno spostamento a livello europeo di una serie di poteri e di competenze di fatto. È certamente un passaggio necessario. Non possono stare in piedi i vincoli e le opportunità di una moneta unica senza un maggiore coordinamento e una maggiore integrazione delle politiche fiscali.

esclusivamente dentro il recinto delle responsabilità della Commissione e dei Capi di Governo; per questo abbiamo chiesto con urgenza questo dibattito. Occorre che un passaggio così impegnativo sia sostenuto da una convinzione nell'opinione pubblica, da una forte base nei Parlamenti nazionali dalla costruzione di una coscienza collettiva dei Paesi. È una realtà che non può essere minimizzata, e trovo singolare l'atteggiamento del Ministro, che comunica all'opinione pubblica che sostanzialmente non cambierà nulla. Cambierà molto, e cercherò di dimostrare quali saranno le conseguenze per l'Italia. Certo, il principio è assolutamente condivisibile. In sostanza, non si può vivere troppo a lungo al di sopra delle proprie possibilità, ma occorre raggiungere un equilibrio. Dunque, se l'obiettivo è del tutto condivisibile, dobbiamo anche riflettere però su alcuni limiti, su alcuni problemi che resteranno aperti. Il primo è evidente: generalizzate politiche di bilancio fortemente restrittive, attuate nello stesso tempo, quali effetti deflazionistici possono comportare? Quindi, c'è il tema dell'equilibrio, che non può essere raggiunto solo attraverso il rigore delle politiche finanziarie: occorre anche un forte impegno per lo sviluppo.

Tuttavia, anche qui dobbiamo riflettere: le sanzioni previste sono veramente molto dure, ed è chiaro che la Commissione punta su un loro effetto dissuasivo (perché poi, se veramente dovessero essere si avrà la possibilità e la forza di imporle?). Se un Governo gioca sull'azzardo - è successo in Grecia - può fallire politicamente, ma poi è credibile che il nuovo Governo possa essere caricato di sanzioni che finiscono per ostacolare una politica di ripresa e di controllo della finanza pubblica? Forse si può puntare un po' di più su sanzioni che riguardano la reputazione di quei Governi, ad esempio intervenendo anche sulle limitazioni del diritto di voto. Terzo aspetto: c'è certamente il rischio di un cortocircuito democratico. Può la tecnocrazia sostituirsi alla politica ed alla rappresentanza democratica? Può un livello che è senza sanzione elettorale applicare e imporre politiche a livelli che sono espressione di una rappresentanza? Infine, ricordiamo che il problema non riguarda solo il debito pubblico. Irlanda e Spagna, ad esempio, nel 2007, prima che iniziasse la grande crisi, avevano un attivo di bilancio rispettivamente dello 0,3 e dell'1,9 per cento e un debito al 25 e al 36 quindi la crisi non nasce da quel difetto di finanza pubblica, ma da una straordinaria espansione del credito che ha creato delle bolle finanziarie e immobiliari che hanno portato questi Paesi in una situazione di difficoltà. Vi è quindi la necessità di integrare maggiormente anche le politiche creditizie e per questo si sono creati gli strumenti del Comitato europeo del rischio sistemico e la nuova autorità di vigilanza bancaria, che certamente potrà offrire delle politiche. Cosa può accadere per l'Italia? Penso che il nostro Paese possa e debba utilizzare questo vincolo esterno per migliorare la sostenibilità della finanza pubblica e le condizioni di competitività del Paese. È successo in passato positivamente: può succedere anche oggi. Le conseguenze ci sono, e sono impegnative. anzitutto quelle formali: naturalmente, la nostra legge di contabilità è del tutto superata da questa nuova programmazione (magari il Governo potrebbe per il momento attenersi a quei vincoli di legge e non immaginare che la legge di stabilità non serva a nulla e che si farà un decreto-legge di fine anno scavalcando ogni procedura). necessità di dotarsi di strumenti adeguati, come prevede il documento della *task* *force*. A livello nazionale la *task force* raccomanda l'uso o la creazione di istituzioni e organismi pubblici in grado di fornire analisi, valutazioni e previsioni indipendenti su questioni di politica fiscale quale strumento per rafforzare la *governance* di bilancio ed assicurare la sostenibilità a lungo termine. Perché il ministro Tremonti, componente della *task force*, firma questo documento ed in Italia non dà retta alle nostre proposte

di un unico Servizio parlamentare del bilancio, dotato di tutte le competenze necessarie? Perché, signora Presidente e signor rappresentante del Governo, questo Ministro, che sottolinea l'importanza del ruolo delle autorità indipendenti,

Certamente è importante per noi che tra gli elementi che verranno considerati ci siano elementi in cui registriamo migliori risultati rispetto ad altri Paesi: pensiamo, ad esempio, al debito del settore privato, al debito verso l'estero, alla quota del settore immobiliare, al sistema bancario. Sono settori in cui stiamo relativamente meglio rispetto ad altri Paesi europei, ma non dimentichiamo che ci sono altri settori in cui stiamo molto peggio: non solo la questione del rapporto debito-PIL, ma le partite correnti, la competitività globale del sistema, la pressione fiscale, la rigidità della spesa.

obbligatorio del 5 per cento annuo sull'eccedenza del livello del debito rispetto al 60 per cento, per noi sarà un percorso molto, molto difficile; ma dipenderà dal livello di crescita.

Se invece la crescita fosse, più realisticamente, pari all'un per cento, cioè se crescessimo di quel tanto che siamo cresciuti negli anni precedenti, al netto degli anni della crisi?

immediatamente il livello del 120 per cento del debito a cui siamo arrivati e solo se riusciamo a correggere la deriva della bassa crescita che renderebbe insostenibile l'impegno che i documenti ci richiedono. Per abbattere il gradino così elevato del debito

del patrimonio pubblico (certo, coraggiosa, e con le difficoltà che ci sono) e di un'iniziativa coraggiosa, chiedendo ai grandi patrimoni privati un intervento *una tantum* che consenta di aggredire questa massa del debito. Ci sono poi anche proposte che andrebbero approfondite circa decisioni a livello sovranazionale: ad esempio, in diverse sedi si è proposta la possibilità di trasferire ad organismi internazionali quote di debito sovrano dei vari Paesi, quindi scorporandole dai bilanci nazionali attraverso la creazione di un fondo

Vi è poi la diminuzione del costo dei fattori. Negli ultimi anni abbiamo molto lavorato sulla diminuzione del costo del lavoro; secondo me c'è stato un eccesso, si è premuto troppo il pedale sul costo del lavoro, producendo un eccesso di precarizzazione con abbassamento dei salari reali. Ci sono altri fattori produttivi su cui intervenire (liberalizzazioni, costo dei servizi, logistica, energia), rispetto ai quali la mozione del senatore Rutelli ci dà molti suggerimenti. Resta un intervento che possiamo praticare: un aumento della produttività e della competitività totale dei fattori vuol dire riforme,

l'Italia nell'euro non fu solo per la loro credibilità personale, ma perché il Paese aveva avuto il coraggio di fare una riforma delle pensioni che ha reso credibili gli impegni che poi avremmo assunto con l'entrata nell'euro.

Presidente, depositerò agli atti il mio intervento scritto, ma mi consenta di approfittare di questi pochi minuti semplicemente per fare delle riflessioni che non avevo scritto, ma che derivano dal dibattito che ho ascoltato con molta attenzione questa sera.

corrisponda uguale salario. Mi fermo qui, perché probabilmente dovremmo fare una discussione, visto che abbiamo le idee confuse anche a questo

di un più che sottile, strisciante euroscetticismo, perché l'Europa - e lei che è stata un ottimo commissario europeo, Presidente, lo sa - non è soltanto la Banca centrale europea.

L'Europa vuole invece che i singoli Paesi crescano, tant'è che investe anche su questo. Il fatto è che noi probabilmente abbiamo o scarsa dimestichezza rispetto agli *input* che ci vengono dall'Unione europea, oppure una scarsa valutazione di ciò che l'Europa vuol fare per i singoli Paesi e addirittura per le singole regioni. Persino per l'utilizzo dei fondi strutturali o dei fondi

quelle regioni in ritardo di sviluppo. In questo senso, mi si consenta di fare un'ulteriore riflessione sul dibattito che si è svolto nel

quando ancora il Senato non aveva deciso cosa fare e che indirizzo dare. Oggi sarebbe stato molto più interessante che ci fossimo soffermati di più sui contenuti della mozione del del senatore Rutelli, che erano contenuti di politica economica nazionale, rispetto ai quali non si può prescindere, per andare poi in Europa a raccontare cosa l'Italia vuole fare in termini di politica economica, cosa l'Italia vuole fare per crescere, svilupparsi e non rimanere con l'angoscia ed il problema del debito, dal quale non sa come uscire. Ma noi cosa andiamo a dire in Europa? Anche nel dibattito

Per esempio, ci sarebbe piaciuto questa sera soffermarci di più su quelli che possono essere gli interventi, non assistenziali, ma gli interventi per le famiglie, gli interventi di politica fiscale per aiutare realmente, questo nucleo, che per noi è ancora un nucleo fondante

per dire agli altri cosa effettivamente l'Italia vuole fare. Io sono amareggiata, per quello che può contare la mia amarezza, per questo modo di legiferare e, soprattutto, per questo modo di partecipare al rapporto con l'Europa, che è diventato un rapporto semplicemente formale e burocratico, privo di quell'anima che noi, invece, dovremmo mettere in un rapporto più consapevole e denso di contenuti con la nostra Europa. Probabilmente, o non consideriamo l'Europa o, forse, riteniamo di essere talmente deboli nella contrattazione con l'Europa che non valga neanche la pena di discutere di contenuti.

L'atto di cui parlo riguarda una tematica su cui si è incentrata l'attenzione di settori importanti dell'opinione pubblica, in quanto, per effetto per effetto di una decisione contenuta nel decreto incentivi, chi fosse nella condizione di aver vinto i primi due gradi di giudizio ed avesse controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di cassazione può risolvere il proprio contenzioso pagando il 5 per cento del valore della controversia, con la contestuale rinuncia da parte del fisco ad ogni ulteriore pretesa. Noi sappiamo che di questa norma si è sicuramente avvalsa la società editrice Mondadori, uscendo, con un esborso relativamente contenuto, di 8,6 milioni di euro, da un contenzioso che avrebbe comportato, se l'azienda fosse risultata soccombente in giudizio, una spesa di circa 350 milioni di euro. Ma non sappiamo se la Mondadori è stata l'unica azienda a beneficiare della norma o se altri se ne sono potuti giovare, per quali importi versati, né a quanto ammontino, eventualmente, le somme cui abbia

Ora, signora Presidente, io debbo lamentare, come molti colleghi insistentemente denunciano, la scarsa propensione del Governo, ed è un eufemismo, a rispondere sollecitamente alle interrogazioni che vengono presentate. È, in generale, un segno di arroganza e di supponenza nei confronti del Parlamento e, soprattutto, di svilimento dei diritti dell'opposizione. Nel caso di specie, però, per l'attenzione generale che circonda questa questione, sottrarsi dal dare puntuali riscontri alle domande formulate (visto che i termini per avvalersi di quel beneficio sono scaduti da due mesi e, quindi, non vi è nessuna ragione per avere comportamenti dilatori) è una conferma evidente, se si persiste in questo atteggiamento, d'imbarazzo, che autorizza a dar credito alle interpretazioni più severe e critiche in merito alle discutibili sovrapposizioni d'interessi che coinvolgono, certamente il Presidente del Consiglio, ma anche il ruolo del ministro dell'economia Tremonti.